*(PD)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, signor rappresentante del Governo, intervengo per esprimere un giudizio fortemente critico sul complesso del DPEF, che presenta lacune e contraddizioni inammissibili. dal fatto che non si leggono percorsi, per quanto in fase di programmazione, idonei o indicativi per uscire da una crisi economica che attanaglia il nostro Paese. Anzi, non solo non vengono affrontate le problematiche nella loro complessità, ma il documento appare quanto mai vago ed inconcludente.

Ci si chiede ove sia un qualsiasi riferimento alla tanto declamata centralità del cittadino e a tutte le azioni che ne derivano. Ed allora delle due l'una: o il Libro bianco contiene fandonie o il DPEF è un documento programmatico inadeguato ad affrontare le vere problematiche degli italiani. Il rinnovamento del pubblico impiego non passa per una demonizzazione. Un *welfare* adeguato alle nuove e reali esigenze, un adeguato apporto ai bisogni di una società che si è rinnovata sono problemi di tutti e di cui tutti devono farsi carico, non solo alcuni.

Nel DPEF non ci sono riferimenti programmatici sulla sanità, parte fondamentale e assolutamente legata a tutto il sistema del *welfare*. Non avere idee programmatiche sull'assistenza sanitaria significa svilire non solo uno dei diritti fondamentali della Costituzione, ma anche quelli descritti nello stesso Libro bianco.

Termino evidenziando che il documento parla di potenziamento delle infrastrutture, mentre i tendenziali indicano una caduta di diversi miliardi delle relative risorse. potrei che congratularmi con il Governo se si realizzassero le previsioni contenute sulla lotta all'evasione e sui suoi frutti, sempre messi in conto come ingentissimi, pur constatando che poi purtroppo che la realtà è spesso deludente. Prendo atto che si continua a navigare a vista.

con un bilancio pubblico fuori controllo non credo veramente che si possa stare allegri. Forse, se aveste ascoltato qualche volta anche l'opposizione, e magari il mio partito, queste situazioni non si

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, un anno fa, e con una lungimirante iniziativa del Governo, con il decreto-legge n. 93 del 2008, si provvedeva a mettere in sicurezza i conti pubblici anticipando di fatto una manovra finanziaria che, se rinviata al successivo autunno, avrebbe esposto in misura ben più grave il sistema Italia ai contraccolpi di una profonda crisi internazionale. L'anticipazione delle misure a carattere economico-finanziario è stata una scelta che ha consentito al nostro Paese di affrontare con relativa sicurezza le difficoltà via via emerse.

si pongono le basi per un definitivo superamento della crisi finanziaria internazionale, individuando un percorso che, con ogni probabilità, sarà ancora lungo e faticoso, ma riguardo al quale possiamo senz'altro dire di avere superato il punto più difficile. Il Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 presenta un quadro realistico dell'attuale situazione, illustrando le strategie che il bilancio dello Stato è in grado di attuare per accompagnare il Paese verso una stagione di crescita, ma senza nascondere le difficoltà che ancora ci separano da una situazione di sicurezza, e soprattutto senza tacere la difficile eredità in termini di debito pubblico, che questo passaggio determinerà sui conti dello Stato. L'analisi non può prescindere da un dato di fatto estremamente pesante, ovvero che il 2009 fa segnare la più forte contrazione del commercio mondiale mai registrata nel secondo dopoguerra, quindi nell'arco degli ultimi 60 anni. La riduzione dei traffici internazionali si attesta per l'anno in corso attorno al 16,2 per cento, un dato già preoccupante, a fronte del quale le esportazioni italiane fanno segnare un arretramento del 19,2 per cento, mentre le importazioni subiscono un ridimensionamento del 15,3 Questi numeri confermano quanto abbia pesato sull'Italia, per la rilevanza dell'industria manifatturiera del nostro Paese e per la notevole propensione all'*export*, un crollo di simili dimensioni degli scambi mondiali. Un calo delle esportazioni che sfiora un quinto del totale costituisce un ridimensionamento che non può essere automaticamente colmato da una fase di crescita come si annuncia già a partire dal 2010, in concomitanza con la ripresa degli scambi internazionali. Vale a dire che, dopo un simile sconvolgimento del nostro *export*, non è affatto automatico che la fase di recupero sia tale da riportare tutti i settori, tutte le imprese, alla medesima situazione pre-crisi. Per questo appare estremamente rilevante che, come è avvenuto con il decreto-legge n. 78 che esamineremo (ad esempio, con gli sgravi fiscali per gli investimenti), ci si proietti con notevole anticipo verso la fase della ripresa, in modo da offrire alle aziende italiane gli strumenti per assicurarsi una rinnovata competitività in termini di tecnologia, di innovazione, di *design*, di capacità di interpretare e accompagnare le tendenze del mercato. Il sistema Italia è in grado di cogliere questa sfida, oltre che per le caratteristiche di intraprendenza della nostra imprenditoria e per l'alta professionalità delle risorse umane, anche in ragione di una solidità di base, dovuta all'indebitamento aggregato - pubblica amministrazione, famiglie, imprese - che presenta valori inferiori a quelli di altri Paesi paragonabili al nostro per dimensione e struttura sociale. sociale. Alcuni segnali ci sono già. È da ricordare il significativo rallentamento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte dell'industria nel mese di giugno. Sono segnali un'imminente ripresa, alla quale ha indubbiamente contribuito il pacchetto di stimoli fiscali messo a punto, già alla fine del 2008, dal Governo. Sono stimoli che si basano su quattro assi di intervento: le imprese, il mercato del lavoro, il potere d'acquisto (quindi le famiglie), e le infrastrutture. Oltre agli aiuti monetari sono state messe in atto misure sistematiche volte a ricreare fiducia per le famiglie e per le imprese o indirizzare alla semplificazione e snellimento delle procedure, che non sono facilmente quantificabili, ma che contribuiscono a consolidare il sistema Paese. C'è da auspicare che la prossima ripresa offra l'opportunità, a fronte di una macchina pubblica più efficiente, di ridisegnare in modo sostanziale la destinazione delle risorse.

signor Vice Ministro, il DPEF in discussione, l'ultimo per via della riforma della contabilità già licenziata in Senato, che certamente nessuno rimpiangerà per le sue contraddizioni, contiene, analogamente agli ultimi provvedimenti approvati (quasi sempre a colpi di maggioranza), molto fumo e poco arrosto. Sono le stesse cifre elencate a smontare le propagandistiche misure di sostegno all'economia che lievitavano nei mesi scorsi fino a 80 miliardi di euro ed annunciate nei consessi internazionali in una politica al rialzo, una politica al rialzo, a smontare la propaganda del Governo. Basta leggere l'ultimo rapporto del Fondo monetario: «L'incidenza dei provvedimenti con il sostegno pubblico diretto, in percentuale del del 2008, è risultata maggiore nei Paesi anglosassoni, perché in Italia non vi è stata necessità di intervenire a sostegno del sistema finanziario».

una massiccia perdita di posti di lavoro, stimata dal CNEL (che non è presieduto da quei catastrofisti dell'Italia dei Valori, ma da un ex ministro del Governo Berlusconi, Antonio Marzano) in 500.000 unità, con un tasso di disoccupazione che si potrà collocare all'8,8 per cento

la biblioteca del Senato è stata illustrata dal cardinal Bertone l'enciclica di Benedetto XVI "Caritas in veritate": penso che bisognerebbe seguire quei consigli: «Le autorità pubbliche collocate ai diversi livelli di governo devono consentire, anzi favorire, la nascita e il rafforzamento di un mercato finanziario pluralista, un mercato cioè in cui possano operare in condizioni di oggettiva parità soggetti diversi». È il contrario di quanto state facendo, salvaguardando monopoli e cartelli. Bertone suggerisce anche di pensare «alle banche del territorio (...) enti che non solamente non propongono ai propri sportelli finanza creativa, ma soprattutto svolgono un ruolo complementare, e dunque equilibratore, rispetto agli agenti della finanza speculativa». Se negli ultimi decenni le autorità finanziarie avessero tolto i tanti vincoli che gravano sui soggetti della finanza alternativa, la crisi odierna non avrebbe avuto la potenza devastatrice che stiamo conoscendo. Voi, piuttosto che tagliare le unghie alla cupidigia dei banchieri, alla loro avidità, ci andate a braccetto anche in questo DPEF. Un Governo ed un Ministro dell'economia seri, responsabili ed anche meno tifosi del colbertismo, avevano l'obbligo di ampliare le misure a sostegno dei redditi dei soggetti più deboli, per poter rilanciare i consumi. Spiace rilevare che oltre all'estensione, con successivi atti amministrativi, della "umilia *card*" non troviamo nulla di interessante per rilanciare l'economia ed aiutare soprattutto quel 1.600.000 di lavoratori impoveriti (stimati dalla Banca d'Italia), i quali ci sono tanti lavoratori atipici. L'incidenza della povertà, che è in aumento, è stimata al 47 per cento. Il DPEF tace sullo scudo fiscale, la più grande operazione di riciclaggio di Stato, dove il Ministro colbertista appare un insuperabile maestro nel dirigere la grande lavanderia statale per far ripulire i capitali frutto di attività illecite, attività mafiose o paramafiose dei «furbetti del quartierino», con i quali sembra che andiate a braccetto, come dei grandi evasori. Somme esportate nei paradisi fiscali e negli Stati canaglia, armi e droga, dal contrabbando e da qualsiasi altra attività criminale. Tutto ripulito in forma anonima, a differenza degli altri Paesi. Questo è un Governo che premia gli evasori e i criminali per favorire il rientro dei capitali mafiosi. Per fortuna avete corretto la stangata sui terremotati, perché volevate far pagare le tasse, con tutti gli arretrati, dal 1° gennaio prossimo a chi ha perso la propria abitazione e qualsiasi possibilità di attività produttiva. Nel DPEF tremontian-leghista non esiste alcuna analisi o riferimento agli allarmanti dati che riguardano l'economia meridionale in agonia, come afferma l'ultimo rapporto SVIMEZ: in dieci anni, dal 1997 al 2008, circa 700.000 persone hanno abbandonato il Mezzogiorno, e non si tratta di manovalanza generica. Per fronteggiare i disavanzi dei Comuni di Catania e di Roma il Governo, maturando la convinzione che con il Sud non ci sia più niente da fare, da una parte annuncia la costituzione di una Banca per il Sud, dall'altra ipoteca le risorse pubbliche nazionali per il Sud fino al 2015, sequestrando i fondi FAS con una partita di giro, che potrebbe anche essere definita di "raggiro" per le popolazioni meridionali. Per far riprendere l'economia italiana bisogna aumentare i redditi da lavoro e da pensione, incidere sulla loro defiscalizzazione, perché la loro caduta in questi anni è una delle ragioni più profonde della crisi, oltre alla grande questione ancora aperta, relativa alla redistribuzione del reddito tra le classi sociali. destinare le poche risorse pubbliche alla riconversione ecologica dell'economia investendo sulle energie da fonti rinnovabili; aumentare gli elementi di coesione, invece di tentare di emarginare forze sociali importanti, come prevede l'accordo separato che ha escluso la CGIL; migliorare il *welfare* per evitare l'abbandono alla disperazione di intere fasce della popolazione più debole. Malgrado la palese presa d'atto delle dinamiche recessive in atto, le stime del Governo conservano la tendenza ad edulcorare la realtà dei dati: le misure correttive adottate in funzione anticiclica, contenute entro limiti molto esigui, giustificati dalla preoccupazione per i vincoli di bilancio e di debito, non hanno avuto efficacia nel contrastare la crisi. Che manchi una seria politica economica impostata per creare nuova occupazione e nuove misure per offrire un ruolo alla ricerca, all'innovazione e alla modernizzazione del Paese e che in questi 15 mesi l'Esecutivo abbia fatto un vero gioco delle tre carte non lo diciamo solo noi dell'Italia dei Valori. Ha scritto Eugenio Scalfari domenica 26 luglio: «Sono molti, anzi moltissimi gli italiani che di fronte allo scandalo Berlusconi (...) rispondono: "A noi non importano i suoi vizi, privati o pubblici che siano; a noi importa che governi bene nell'interesse del Paese e dei cittadini". Si può essere d'accordo o no su questo modo di ragionare, ma anche se ci adattiamo a questa diffusa indifferenza morale e seguiamo pure quel modo di ragionare, si sta governando bene? Il Governo ha varato un nuovo decreto-legge per contenere la crisi, un decreto pasticciato, come scrivono anche i giornali di oggi. Si susseguono un pasticcio dietro l'altro: dietro l'altro: bisogna varare decreti correttivi di decreti che ancora devono essere approvati! visto, è arrivato al 5,2 del PIL ed è molto probabile che salga ancora. In parte questo pessimo risultato è dovuto a cause internazionali, ma in altra parte è dovuto a cause esclusivamente interne, e cioè all'andamento della spesa pubblica e delle entrate. La spesa è aumentata in un anno del 4,9 per cento: in cifre assolute si tratta di 35 miliardi di euro. Stiamo parlando di spesa corrente della pubblica amministrazione. Come è stato possibile uno sfondamento di queste dimensioni, che equivale ad una buona manovra finanziaria? Questo dato mette in evidenza una non prevista espansione della spesa ordinaria della pubblica amministrazione di fronte ad una preoccupante caduta degli investimenti. Tutto ciò, in presenza di una diminuzione del peso degli interessi sul debito pubblico per effetto della caduta dei tassi Questi tassi di interesse, come ha detto anche il relatore, sono destinati ad aumentare; quindi, bisogna mettere in

Si può anche comprendere che il *Premier* non voglia rispondere sulle veline e sulle *escort*, e noi dell'Italia dei Valori abbiamo ripugnato la politica che scruta dal buco della serratura, ma qui stiamo ponendo una domanda di tutt'altra natura: signor Vice Ministro, che cosa ne avete fatto di quei 35 miliardi di maggiori spese in un anno di vacche magrissime? Ci potreste rispondere che quei miliardi li avete usati per "stimolare" l'economia, invece neppure quello avete fatto. I denari freschi per stimolare o sostenere l'economia ammontano, in tutto e per tutto, a 3 miliardi di euro, pari allo 0,2 per cento del prodotto nazionale lordo

la caduta del prezzo degli immobili, eppure prevedete di continuare a saccheggiare il territorio, le coste, l'ambiente, l'ambiente, e di continuare a costruire alloggi. I progetti saranno certificati da un professionista di fiducia del committente. Sono veramente necessarie queste case, con le quali il territorio sarà definitivamente devastato? Un altro esempio, signori rappresentanti del Governo, riguarda la messa sotto schiaffo, con il cosiddetto lodo Bernardo, della Corte dei conti, che il Governo sta riducendo a un simulacro, manomettendo i suoi poteri di controllo sulla pubblica amministrazione. Anche su questo dovete fare un'indecorosa marcia indietro. Concludo, signor Presidente, per criticare un DPEF sbagliato, frutto di una politica economica errata e fraudolenta nei confronti dei diritti e degli interessi dei cittadini, delle piccole e medie imprese e delle famiglie, che invece di stimolare i consumi affossa la domanda per elargire qualche piccola prebenda in cambio di un consenso che viaggia su un piano inclinato e che marca la distanza dal Paese reale e dalle angosce della povera gente, che fa sempre più fatica per sopravvivere.

sebbene abbia superato la sua fase più acuta, necessita, per essere definitivamente lasciata alle spalle, di interventi programmati su un arco temporale di medio periodo e mirati in funzione di un numero di obiettivi limitato, ma di rilevanza strategica. Il Governo ha, fino ad oggi, brillantemente risposto a questa esigenza mettendo a punto e realizzando una serie continua di interventi che, nel loro insieme, hanno dato luogo a misure flessibili ed efficaci, con le quali è stata data una risposta seria e concreta ai problemi posti dalla crisi in atto. Il Documento di programmazione economico-finanziaria costituisce, come noto, il momento più qualificante ai fini della definizione degli obiettivi e degli strumenti per la politica economica del nostro Paese. La politica economica, oltre che per le misure di carattere generale, si caratterizza per l'articolazione settoriale degli interventi, attraverso la quale è possibile comprendere quali siano le leve strategiche su cui si intende intervenire, al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico del nostro Paese e del nostro territorio. In tutto questo, l'importanza del settore agricolo è, come noto, da misurarsi non solo in riferimento ai suoi valori produttivi, ma anche e soprattutto per il ruolo che lo stesso settore svolge su tutto il territorio nazionale e quindi in relazione alle numerose funzioni di interesse collettivo che esso riveste che esso riveste e assolve in favore della nostra società. È pertanto indispensabile che una politica economica impostata in funzione delle effettive esigenze di sviluppo del nostro sistema socio-economico valorizzi il ruolo strategico del nostro mondo agricolo, considerando la politica agraria come una componente fondamentale dell'economia generale del nostro Paese. Il Governo, anche in questa circostanza, ha evidenziato un'attenzione particolare nel riservare i giusti spazi alle misure di politica agraria che dovranno essere sostenute nell'ambito della politica economica che si intende attuare nel nostro Paese per i prossimi anni. Ciò risulta chiaramente dagli obiettivi e dagli strumenti indicati nella parte agricola del DPEF. Obiettivi e strumenti che sono da considerare decisamente coerenti sia con la generale necessità di sostenere lo sviluppo economico al fine di superare la crisi, sia con le potenzialità e le esigenze di sviluppo della nostra agricoltura. In particolare, per quanto attiene agli obiettivi, riteniamo che lo sviluppo della competitività del settore, la difesa del*made in Italy* e il potenziamento delle infrastrutture rispondano pienamente alle esigenze di un settore che, specie in questa fase di difficoltà, ha in primo luogo la necessità di accrescere il proprio peso contrattuale all'interno delle filiere agroalimentari, dove attualmente il reddito degli agricoltori è fortemente penalizzato. Dobbiamo riflettere sul fatto che - cito un esempio lampante - per ogni euro di spesa solo 17 centesimi vanno a remunerare la fase agricola 60 centesimi vanno alla distribuzione e 23 centesimi vanno all'industria), determinando un progressivo impoverimento ed indebolimento del nostro settore agricolo. Dobbiamo quindi tutelare e valorizzare le nostre produzioni sui mercati esteri, dove il problema della contraffazione e dell'agro-pirateria ha raggiunto livelli preoccupanti, facendo segnare un volume di affari di circa 50 miliardi di euro, addirittura superiore al valore della nostra produzione agricola nazionale. Dobbiamo superare antichi*deficit* strutturali, legati anche alle carenze infrastrutturali e, tra queste, ai problemi legati alla gestione delle risorse idriche (antico problema del nostro Paese). In questo DPEF il Governo ha dimostrato particolare attenzione al mondo agricolo, predisponendo un piano finanziario cospicuo, sicuramente corposo e particolarmente adeguato alle esigenze del momento. In particolare, ai fini dello sviluppo della competitività delle imprese, si punta ad interventi sul fronte delle agevolazioni e, in specie, sul potenziamento delle dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale (anche al fine di colmare le gravi carenze finanziarie degli anni scorsi), e sulla stabilizzazione, in misure a regime, sia delle agevolazioni previdenziali per le aree svantaggiate, sia dell'azzeramento delle accise sul gasolio per le coltivazioni sotto serra. È strategicamente importante la difesa del *made* *in* *Italy*, dove si intende proseguire sulla via, già decisamente intrapresa, del rafforzamento delle strutture deputate ai controlli e del rilancio dell'azienda Buonitalia, al fine di sostenere la promozione dell'agroalimentare e l'internazionalizzazione delle imprese. Concludendo, ritengo che sia rilevante il potenziamento delle infrastrutture, dove si prevede di concentrare gli sforzi sulle opere irrigue, attraverso il ripristino degli stanziamenti che già erano stati fissati precedentemente per l'attuazione del piano irriguo nazionale. Si tratta di un impegno programmatico importante, che trova effettivo riscontro nel volume delle risorse che si intendono mobilitare in favore del settore agricolo, verso il quale saranno stanziati ben 793 milioni di euro.

*green* *economy*. Questo è molto grave, per due ragioni. In primo luogo, perché la prospettiva dell'economia verde, e delle politiche pubbliche necessarie per realizzarla e concretizzarla, ha un grande rilievo in considerazione della necessità di fronteggiare la crisi economica (quindi nel breve

nel G8, e ancora prima con il pacchetto clima, e che sta per assumere, presumibilmente in occasione della Conferenza di Copenaghen del prossimo dicembre riguardo alla minaccia globale rappresentata dai cambiamenti climatici. Nella stragrande maggioranza dei Paesi industrializzati i piani di fronteggiamento e di stimolo anticiclico contro la crisi comprendono in modo sostanziale incentivi, misure fiscali ed investimenti pubblici rivolti a stimolare la *green economy*. In Italia di tutto ciò non c'è traccia, e questo vale Le misure su cui possiamo contare sono state quasi sempre adottate dagli ultimi Governi di centrosinistra, mentre l'attuale Governo, in più di un'occasione, ha addirittura varato provvedimenti che penalizzano lo sforzo di innovazione. L'ultimo caso è il disegno di legge su energia e sviluppo, appena approvato, che prevede l'obbligo per i piccoli impianti di cogenerazione non allacciati alla rete elettrica di pagare comunque gli oneri di dispacciamento, largamente sottofinanziati capitoli decisivi: penso alle bonifiche, alla mobilità sostenibile, all'implementazione di nuove legislazioni comunitarie come

*(PD)*. Signor Presidente, signori del Governo, intervengo innanzitutto per sottolineare che anche in questa occasione la tempistica viene largamente disattesa, impedendo così al Parlamento di procedere a un esame approfondito di un provvedimento, qual è il Documento di programmazione economico-finanziaria, vincolante per le decisioni successive. Siamo quindi in presenza dell'ennesima violazione delle prerogative del Parlamento, che non può essere taciuta e che ormai rappresenta una costante dell'attività legislativa del Governo. Per venire al merito presenta un Documento di programmazione economico-finanziaria che, da una parte, afferma che siamo di fronte alla crisi economica più grave dal secondo dopoguerra e, dall'altra, sostiene che durante la crisi come se essa fosse ormai passata - ha agito in modo mirato, attraverso una pluralità di interventi, per garantire la stabilità della finanza pubblica, per supportare l'economia e per assicurare la coesione sociale.

quali sarebbero i risultati di una serie di interventi, l'ultimo dei quali - ma sarebbe più corretto dire il penultimo - approderà in quest'Aula nei prossimi giorni? Insisto, quali sarebbero questi risultati? Se guardo ai dati sull'andamento dell'economia e le previsioni contenute nel DPEF, vedo una situazione completamente diversa da quella che voi raccontate

una riduzione della produzione industriale del 27 per cento, un calo degli ordinativi del 30 per cento e una caduta delle esportazioni del 30 economico-finanziaria - quindi non altre fonti - prevede un calo del PIL del 5,2 per cento, un debito pubblico che sfiora ormai il 120 per cento. Infatti, calano le entrate e aumentano in maniera paurosa le spese; chi ha fatto i conti parla di 35 miliardi di aumento della spesa primaria. Inoltre, la previsione sull'occupazione è davvero preoccupante perché il tasso di disoccupazione viaggia ormai verso il 10 non a caso nei giorni scorsi ha parlato di 500.000 posti di lavoro a rischio per il 2009. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria si afferma però che negli ultimi due, tre mesi si sono ripetuti segnali non negativi, ma nello stesso Documento, subito dopo, si sostiene che la previsione di ripresa per il 2010 è sostanzialmente vicina allo zero: è previsto un aumento del prodotto

perché segnala che la ripresa economica nei prossimi anni sarà comunque molto lenta e che per il nostro Paese sarà ancora più difficoltosa

di questo drammatico problema sociale che il Documento di programmazione economico-finanziaria mostra tutta la sua inadeguatezza e la sua mancanza di visione programmatica. Infatti, non solo non prevede alcuna riduzione fiscale per i redditi da lavoro e da pensione quindi, indirettamente, nessun sostegno al rilancio dei consumi ma, soprattutto, rinvia ancora la riforma degli ammortizzatori sociali, lasciando così i lavoratori precari e delle piccole aziende senza tutele. In sostanza, per concludere, è un DPEF assolutamente inadeguato sul versante economico e sociale e totalmente incapace di governare il debito pubblico. Sentiremo poi il ministro Tremonti, al quale in particolare mi riferisco, ma altro che coesione sociale: dopo i condoni ci aspettano i tagli alle pensioni e alla sanità e questo indubbiamente alimenterà nuove tensioni sociali che metteranno a dura prova la tenuta economica del Paese.

è giunto all'attenzione, non solo mediatica, ma anche del Governo e del Parlamento. Il problema è che vi è giunto nel modo peggiore: non per un confronto che si sviluppa su proposte che non vi sono,

dibattiti extraistituzionali, ma ascoltare il sottosegretario Bonaiuti, ineffabile nel considerare che il tema del Mezzogiorno non esiste che è soltanto una enfatizzazione mediatica perché davvero il Governo fino ad oggi ha fatto tanto per il Sud, mi preoccupa. Vuol dire, infatti, la consapevolezza delle difficoltà non è patrimonio del Governo, o comunque di espressioni autorevoli del Governo, e che, quindi, io devo immaginare che le rassicurazioni del Presidente del Consiglio su una strategia importante ed innovativa, volta ad innescare processi di sviluppo nel Sud, siano un annuncio come altri che poi non raggiungono sostanza concreta. è una conferma alle mie preoccupazioni. Questo documento, cui avete dato un'impostazione minimalista, una sorta di obbligo formale cui ottemperare perché in altri provvedimenti si sviluppa l'azione di governo,

che questo documento possa costituire ancora un elemento essenziale per un corretto e trasparente processo di programmazione economica in quanto, premettendo la valutazione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati, stabilisce gli obiettivi fondamentali della politica economica per il periodo di riferimento. A legislazione vigente, la sessione di bilancio ha regole ben precise nei tempi e nei modi. di programmazione economico-finanziaria mediante risoluzioni con cui si stabiliscono le entità della manovra nonché le cifre e le modalità attraverso cui questa entità verrà indicata nei saldi di finanza pubblica non rappresenta un atto rappresenta un atto formale a carattere meramente programmatico, ma costituisce l'atto attraverso cui Parlamento e Governo sono chiamati ad assumere concordemente decisioni vincolanti per la successiva fase di bilancio nella quale il procedimento legislativo di esame del disegno di legge finanziaria e di bilancio dovrà svilupparsi in modo coerente con le previsioni del DPEF. Come Come già lo scorso anno, anche stavolta la tempistica viene invertita. È la manovra che anticipa e vincola il Documento ci fu spiegato che rispetto alla drammaticità della crisi e alle sue ripercussioni sulla stabilità della nostra finanza pubblica occorreva mettere in sicurezza il bilancio dello Stato e procedere con misure drastiche che invertivano anche la tempistica dei documenti finanziari. Questo accadeva l'anno scorso. Quest'anno, caro ministro Vegas, vi è stato tutto il tempo di immaginare un corretto dispiegarsi dell'azione di programmazione e di intervento finanziario da parte del Governo

relativamente ad alcuni interventi con i quali il Governo ha cercato di salvaguardare il sistema creditizio, stimolato i consumi, potenziato il sostegno al reddito ed integrato il sistema degli ammortizzatori sociali. anche utilizzando la solidarietà delle Regioni, che hanno reso disponibili risorse importanti per questo strumento essenziale di garanzia in una fase di crisi, lasciando da parte valutazioni sulla ricaduta di tali risorse, perché la gran parte del sistema produttivo, dove questi ammortizzatori sociali esercitano i loro benefici effetti, è allocata in una certa area del Paese. In altre aree quei meccanismi, per la precarietà di quell'economia e di tanti e di tanti rapporti di lavoro che non sono coperti da quegli interventi, non hanno ricadute. Vi era un discorso di solidarietà e di investimento strategico nella garanzia dei livelli occupazionali che rappresenta un interesse nazionale. A questo hanno compartecipato con convinzione le Regioni e in particolare quelle del Mezzogiorno. Lo stesso sforzo

del Sud del Paese e gli impegni che la coalizione aveva assunto in modo solenne attraverso un documento programmatico, che prevedeva come linea strategica essenziale del Governo il recupero del divario attraverso un programma di interventi infrastrutturali e di stimolo all'economia. in discussione che le condizioni di debolezza del meridione del Paese determinano, oltre che la sofferenza di quei territori, anche un indebolimento complessivo della struttura economica nazionale ed un'incapacità a competere del nostro Paese all'interno del sistema europeo.

la scelta precisa del Governo di utilizzare le risorse 2007-2013 programmate

non erano oggetto di programmazione delle amministrazioni regionali ma erano una parte di competenza nazionale che toccava a voi spendere, sulla base di una razionale programmazione ed attraverso l'utilizzo di quel criterio di discernimento, fissato per legge e violato per legge, dell'85

delle classi dirigenti meridionali, su cui grava un giudizio, spesso fondato, di inefficienza, di sperpero e di clientelismo, che serve come alibi per questa operazione di sottrazione

lo Stato dovrebbe predisporre su tutto il suo territorio nazionale.

parlo della Sicilia in modo particolare - si scopre che tutti gli interventi di cui menano vanto l'ANAS e le Ferrovie sono finanziati con fondi europei o fondi FAS,

e puntualmente faremo circolare una nota da cui si possono rilevare tali dati. Gli interventi aggiuntivi divengono sostitutivi e quelli sostitutivi vengono sostituiti ulteriormente, perché spostati da un'altra parte in quanto non vengono attribuiti ai territori che

di modifica delle procedure nell'ambito del CIPE ed anche attraverso posizioni di contestazione sulla programmazione regionale

Ciò che può fare Roma non può fare a Palermo, ma abbiamo accettato anche questo. Abbiamo rivisto il PAR della nostra Regione impegnandolo integralmente per spese in investimenti. Si attende che quelle risorse, ove realmente sopravvissute alla spoliazione, vengano attribuite con celerità, perché la crisi è tale ovunque. Ora, se quest'ultima autorizza il Governo ad invertire la tempistica parlamentare e a razionalità dei documenti finanziari modificando tutte le linee di intervento sul terreno economico, anche

non preoccuparsi perché è un'esigenza contabile temporanea che sarà

conclusa l'opera di requisizione delle risorse assegnate e non spese dei fondi FAS e dei fondi europei

utilizzata per ripristinare quei finanziamenti alla viabilità in Sicilia e Calabria oltre che finanziare la quota FINTECNA per il ponte sullo Stretto. Il finanziamento per il ponte sullo Stretto c'è stato in forma ad oggi insufficiente; delle risorse per la viabilità in Sicilia e Calabria non abbiamo avuto traccia, ma il *leitmotiv* di questo atteggiamento è di rassicurare che alla fine della fiera i conti sarebbero tornati. Sono convinto che la fine della fiera sarà tra cinque anni perché questo è un Governo solido e forte con una grande maggioranza nel Paese, ma i conti vogliamo che comincino a tornare da adesso. quindi smesso di dare deleghe in bianco, per quel poco che la nostra presenza parlamentare potrà consentirci. Da questo momento, quindi, basta con rassicurazioni verbali, ordini del giorno che non impegnano nessuno

Gli imprenditori la accolgono con favore, ma non contiene alcun elemento in linea in linea con lo spirito e l'impegno del recupero del divario perché fotografa la realtà esistente e garantisce la sostanza dell'apparato produttivo di questo Paese. Noi siamo per la fiscalità di vantaggio che elimina l'intermediazione e le burocrazie e garantisce stimoli allo sviluppo. Ci saremmo accontentati, quantomeno per una coerenza formale con l'impegno programmatico, se il cosiddetto Tremonti-*ter* avesse contenuto un differenziale per le imprese del Sud

che contiene una serie di impegni programmatici, perché noi crediamo al valore politico di questo Documento di programmazione. Se alcuni elementi essenziali

di fare risoluzioni a pezzi e, quindi, mio malgrado, sono costretto a mantenere il favore del Governo esclusivamente su una risoluzione per i meccanismi di votazione consuetudinariamente vigenti in Parlamento e, quindi, a dare l'appoggio alla sola proposta Da questo momento decorrono i 30 minuti a disposizione dei Gruppi per avanzare proposte emendative sul testo della proposta di risoluzione n. 4.

onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in questo intervento sulla presentazione del DPEF al Senato cercherò di segnalare, posto il breve tempo concesso, le questioni inerenti la pianificazione infrastrutturale con particolare riferimento al tradizionale allegato infrastrutture. La prima considerazione è se, alla luce del prodotto che viene offerto quest'anno alla nostra discussione, questo può considerarsi ancora un documento di qualche utilità. Lo dico non per pura polemica ma in ragione di due considerazioni: la trasparenza e l'obiettività, caratteristiche che in teoria dovrebbero presiedere all'impostazione di un simile documento. L'una e l'altra caratteristica sembrano invece essere decisamente venute meno. A chi può interessare allora un documento che, anziché rappresentare una sorta di portolano con cui orientarsi nell'intricato e complesso settore delle infrastrutture, costituisce invece l'occasione di un manifesto politico, per giunta mal scritto? Ho trovato singolare il tono e il contenuto del documento fin dalle quattro paginette contenute in premessa, come da tradizione, a firma del Ministro delle infrastrutture. Cito testualmente il passo di apertura: «dal 1980 fino al 2001, cioè, in venti anni, nel nostro Paese gli investimenti infrastrutturali (...) non avevano superato i 14 miliardi dal 2002 ad oggi, in soli cinque anni - cinque e non sette anni perché durante la passata legislatura c'è stato un blocco di tutti gli interventi - siamo riusciti ad appaltare e a cantierare opere per circa 49 miliardi Non credo ci sia bisogno di commentare l'attendibilità di queste affermazioni. E tutto ciò in barba al fatto che, come invece sappiamo benissimo, in questo documento persiste ancora (come ci ricordava «Il Sole 24 Ore» di qualche giorno fa) una straordinaria confusione tra risorse in competenza e risorse di cassa, la cui effettiva spendibilità per i prossimi anni sembra essere davvero risibile. Altro che manovra anticiclica! Sempre nelle quattro paginette, innumerevoli sono poi le volte in cui si articola il ragionamento, partendo da risposte a presunte critiche che, peraltro, nessuno ha formulato, probabilmente nell'affannoso tentativo di ribaltare i termini di questioni che evidentemente si avvertono ormai diffuse nell'opinione pubblica. Capisco le difficoltà e i problemi che il Ministro si è trovato e si trova a fronteggiare, specie all'interno della sua compagine governativa, e in particolare con il Ministro dell'economia, che è sempre più il vero *dominus* di questo Governo e che di fatto ci fa assistere per la prima volta, credo nella storia repubblicana, a un Ministro delle infrastrutture senza portafoglio. Il punto però è un altro: non si può utilizzare un documento istituzionale, e segnatamente un Documento di programmazione economico-finanziaria, a proprio uso e consumo. In ogni documento di pianificazione il Governo dovrebbe essere chiamato a mettere nero su bianco, possibilmente con la massima oggettività, ciò che ha fatto e ciò che intende fare in ragione delle risorse disponibili e di quelle che intende mettere a disposizione. Non dovrebbe essere l'occasione, come invece è, per manifestare soltanto propositi e buone intenzioni, per tutta la parte relativa alle prospettive di sviluppo infrastrutturale del Paese, dalla portualità al trasporto aereo o a quello ferroviario o autostradale. Significativa, in questo senso, la scomparsa degli 800 milioni di euro per gli investimenti sulla banda larga, cosa peraltro da noi temuta da tempo e denunciata con ampio anticipo. La cito perché è la testimonianza plastica di un Governo che, al di là degli annunci e dei proclami, in realtà ha definitivamente abbandonato un progetto organico, ma direi anche solo un progetto, di modernità del Paese, per proporne uno mediatico e assolutamente finto. Eppure, in questa particolare situazione economica, gli investimenti legati alle infrastrutture materiali e immateriali e alle grandi opere pubbliche attese per il rilancio del Paese avrebbero potuto davvero costituire il volano virtuoso dell'azione di Governo nell'affrontare una crisi di proporzioni davvero rilevanti per intensità e durata. Invece questo Governo, dall'esplosione della crisi, si è come seduto sulle sue debolezze e sulle sue fragilità, nonostante la retorica da regime con la relativa e ossequiosa propaganda, fino alla tracotanza ostentata dei suoi numeri in Parlamento di cui dispone acriticamente a proprio piacimento. È come in attesa che la crisi passi insieme alla nottata! Ma così facendo si assume la responsabilità, ogni giorno che passa, di vanificare l'opportunità di trasformazione, di quei cambiamenti necessari che sono sempre insiti in ogni crisi. Insomma, un Governo che, anziché investire sul futuro del Paese scommettendo sull'intrapresa privata, consente l'acquisizione di monopoli pubblici da parte di grandi gruppi privati, favorendo la rendita e la speculazione fondiaria. Un Governo che, così facendo, abbandona, ogni giorno che passa, il rilancio di una seria politica industriale del sistema Paese, accompagnandone, anziché l'uscita dalla crisi e il suo rilancio, il suo mesto declino.

Purtroppo il Mezzogiorno è ancora la vittima sacrificale; non è bastato neanche il sollevamento all'interno dei partiti della maggioranza, nello strano tentativo di proporre partiti del Sud e di sollecitare il Governo perché ponesse attenzione sul tema.

non potendo competere - così come non compete - sul piano economico e produttivo con il Nord, sarebbe complicato se si attivasse una competizione sul piano politico-partitico; anzi sarebbe addirittura una nuova linfa per

Ma la cosa più interessante è quanto questo DPEF dice sulle politiche agrarie del Paese. È interessante perché, non dicendo niente, per lo meno non ci ricorda quanto sta succedendo, o almeno non ricorda al Parlamento che, negli ultimi mesi - e forse anche negli ultimi due anni - c'è un'inversione totale delle politiche agrarie del Paese,

più importante dal punto di vista della penalizzazione alle politiche agrarie del Mezzogiorno. Non sarà sfuggito a chi segue con attenzione le politiche dell'agricoltura siciliana che ormai i prodotti tradizionali dell'agricoltura mediterranea sono praticamente sull'orlo del collasso. Se qualcuno è interessato, basta vedere che cosa è oggi il costo del frumento per

vite, dell'olio e di altri prodotti del Mezzogiorno.

Se poi guardiamo alle politiche dei trasporti c'è soltanto da inorridire: se qualcuno di voi scegliesse quest'anno di farsi una vacanza in Sicilia, si renderebbe conto di dover essere molto attento nel nel prenotare viaggi, soprattutto con le navi o con gli aliscafi, perché oltre il 50 per cento dei collegamenti con le Isole è stato tagliato da questo Governo.

Le Ferrovie annunciano con grande enfasi la Frecciarossa sul collegamento Milano-Roma, ma nulla dicono

Sul piano degli interventi autostradali, le uniche risorse che abbiamo potuto utilizzare erano quelle dei fondi FAS del passato (quelli che, quando c'erano, ci venivano dati e non venivano portati altrove), per costruire le poche autostrade che siamo riusciti che siamo riusciti a realizzare. C'è una situazione di collegamento, soprattutto ferroviario, che è esattamente quella che ci hanno lasciato i Borboni: non ci sono linee ferroviarie nuove.

un indicatore che desse conto della produttività e soprattutto del benessere del Paese era il consumo dei carboidrati:

quando, nella migliore delle ipotesi, ignora alcuni settori produttivi collegati allo sviluppo del Mezzogiorno e, se parla di di settori che potrebbero essere utili al Mezzogiorno, non lo fa certamente in termini di prospettive positive, ma in termini negativi. A prescindere

come ho detto, l'intervento perequativo all'incontrario. Ci auguriamo che almeno nella legge finanziaria i temi che qui vengono ignorati possano essere ripresi e ci si ricordi che c'è una parte del Paese che vuole essere presa in considerazione in termini produttivi e non assistenziali, ma che ha bisogno certamente di un'attenzione particolare.

di risoluzione presentata dalla Lega Nord, tra gli obiettivi primari dell'azione di Governo, in una visione di politica generale nell'interesse della comunità internazionale, c'è anche la tutela del *made in Italy*. La nostra proposta chiede infatti un maggior impegno per la tutela del *made in Italy*, con interventi diretti anche nei confronti dell'Unione europea, affinché vinca il «fare impresa», nel rispetto dei lavoratori,

il blocco dell'economia reale e la conseguente diminuzione delle entrate dello Stato. Come andare incontro a questa crisi, per sconfiggerla?

che possono essere mandati per cercare di risollevare una situazione di produzione oggi in difficoltà - agire per riconoscere e dare a Cesare quel che è di Cesare.

Questa volta l'andamento del *deficit* e la caduta del PIL sono esattamente quelli anticipati dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dall'OCSE, dalla Commissione di Bruxelles, e il ministro Tremonti non può più parlare di congetture inutilmente allarmistiche. Il quadro è completato dall'avanzo primario, che fotografa il saldo di bilancio al netto della spesa per interessi e che torna a collocarsi per la prima volta sotto lo zero, e dalla crescita del debito, che arriverà a sfiorare il prossimo anno il 120 per Allora qual è il punto da cui partire? La vera sorpresa, in questo DPEF, non è tanto nella conferma delle previsioni, che dopo mesi di confusione, di incertezze e di negazioni all'insegna di un ottimismo di maniera, sono finalmente sovrapponibili a quelle predisposte dai maggiori organismi internazionali, quanto piuttosto nello scoprire un'altra conferma. Il Governo, pur riconoscendo che stiamo attraversando uno dei peggiori anni della nostra storia e che gli unici segnali positivi indicati come premonitori di una ripresa sono semplicemente quelli legati a una riduzione della velocità di caduta, di caduta, non intende dare sostanza ad alcun cambiamento di rotta della sua politica economica. Questo paradosso appare del tutto evidente se leggiamo attentamente il quadro di finanza pubblica notiamo come lo scenario naturale - con linguaggio tecnico definito scenario tendenziale - è del tutto analogo allo scenario programmatico, quello che risente degli interventi discrezionali di politica economica che un Governo che ha responsabilità - quando ha responsabilità - dovrebbe assumere. Questo è il vero e significativo nodo centrale del problema, perché questa scelta, definita prudenziale secondo la maggioranza, rinunciataria e pericolosa secondo noi, comporta alcune importantissime conseguenze, che tracciano le specificità di questo DPEF. La prima conseguenza certamente è dal lato della spesa pubblica. Per rendersene conto, basta pensare a un dato: il totale delle spese pubbliche nel 2010 arriverà al 52 per cento del PIL, mentre lo scorso anno era fermo al 49 per cento. In parole semplici, alla fine della grande recessione ci troveremo con una presenza dello Stato nell'economia italiana ben più importante di quella che avevamo prima. E la differenza non sarà dovuta a nuovi programmi infrastrutturali o ad interventi anticiclici, di cui il Paese ha bisogno: dei quasi 23 miliardi di aumento della spesa corrente, solo 3 derivano da interventi anticrisi; tutto il resto è conseguenza in parte della spesa pensionistica e, soprattutto, di una nuova impennata per acquisti di beni e servizi. Così come la spesa in conto capitale subisce un aumento puramente contabile, determinato in larga sostanza dalla necessità del Governo di rilevare gli immobili inseriti nei programmi SCIP. Si chiude così un'altra operazione fallimentare, targata dall'inizio alla fine dall'attuale Ministro dell'economia, di cui sono in pochi a parlare, che presenta un saldo passivo di 1,7 miliardi di euro (che ha peggiorato ulteriormente i conti pubblici) non ha portato alcun guadagno ai cittadini, ma un enorme guadagno agli altri soggetti coinvolti: le banche, gli investitori finanziari, gli immobiliaristi. In sostanza e in soldini, il Governo ha impegnato risorse finanziarie per affrontare la crisi pari allo 0,6 per cento solo con l'ultimo decreto, che era stato annunciato e presentato come la chiave di svolta per imprimere un nuovo slancio alla nostra economia. Ma c'è un'altra importante conseguenza che viene certificata in questo DPEF, ed è che questa crisi globale, quando finirà, ci lascerà in eredità un debito pubblico enorme. questo vale per tutti i Paesi, ma vale ancora di più per l'Italia che, diversamente da altri, ha usato poco ha usato poco o niente il bilancio pubblico, soprattutto per scelta, più ancora che per necessità (come si è voluto far credere), e non ha messo in campo piani di stimolo e di sostegno significativi e, soprattutto, tempestivi. E quando il debito pubblico comincerà a scendere, a partire dal 2013, ci troveremo con gli stessi livelli di debito degli anni '90, di prima che ebbe inizio quella grande opera di risanamento che ci portò nell'euro. Questo è un altro dato che fa seriamente riflettere:

i problemi strutturali del Paese alla fine sono rimasti sempre gli stessi. In questo DPEF ci sono anche altri numeri che fanno paura. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,4 per cento: lo stesso picco storico che toccò nel 1997, l'anno dell'eurotassa, e più di quanto raggiunto nel 2007, anno del tanto vituperato Governo Prodi/Padoa-Schioppa. Il ministro Tremonti ci ha assicurato che le entrate tributarie tengono. Purtroppo, anche in questo caso la realtà è diversa da come la si vuole rappresentare: nel primo trimestre l'IVA è crollata del 10 per cento, mentre nello stesso periodo i consumi sono scesi solo del 2,6 Come si spiega questa differenza? Il Governo lo ha spiegato con un linguaggio tecnico e ci dice che: «una parte del divario sembrerebbe riconducibile ad una ricomposizione dei consumi verso beni essenziali, caratterizzati da aliquote basse». Noi lo traduciamo in «dipietrese», nel linguaggio della gente comune, di quei 20 milioni di italiani, soprattutto lavoratori dipendenti, che pagano le tasse sino all'ultimo centesimo e che ora vedono arrivare l'ennesimo condono per i capitali esportati illegalmente e di cui nel DPEF non si ha il coraggio di parlare né in termini di cassa, né in termini di etica politica. Il divario si spiega con il dilagare dell'evasione,

per una seria riduzione delle imposte (per la quale, ironia della sorte, il centrodestra ha vinto tre elezioni promettendo meno tasse per tutti), ma anche per una seria iniziativa di riduzione delle disuguaglianze sociali. E che siano numeri seri, numeri che producono danni determinando una contribuzione fiscale più alta e creando una concausa dei tagli indiscriminati alla spesa pubblica (quei tagli lineari che non producono riqualificazione della spesa, ma riduzione della qualità dei servizi a scapito delle fasce sociali deboli), se ne è accorto - meglio tardi che mai - anche il presidente della Camera Fini, intervenendo una settimana fa alla presentazione del documento della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ha chiesto maggiori controlli e rivolto un appello a fare di più per il recupero del gettito. Appare chiaro, allora, che la logica del DPEF è molto semplice: si predicano gli obiettivi altisonanti che il Governo aveva proposto e confermato, cioè la stabilità dei conti pubblici, la coesione sociale, la tutela del credito e della liquidità alle imprese, e poi si fa finta di attuare, con norme vuote e risposte truccate, si sceglie di non agire, ci si ferma, a volte si fa marcia indietro, mascherando l'incapacità di prendere una strada sino in fondo, sino a risultati veri e concreti. di risoluzione presentata dal Gruppo dell'Italia dei Valori, molti degli argomenti sono già stati affrontati nel corso della discussione in Aula e dei lavori in Commissione. Non torneremo quindi su diversi di essi, non perché siano più secondari o marginali rispetto ad altri, ma perché riteniamo più utile concentrarsi sul problema vero del DPEF: un Documento che, per legge dello Stato, avrebbe dovuto contenere un'articolazione degli interventi, anche di settore, con la valutazione di massima dell'effetto attribuito a ciascun tipo di intervento e che, al contrario, nel migliore dei casi, è un'opera incompiuta, e nel peggiore dimostra tutta la sua inadeguatezza rispetto ai problemi del nostro Paese. La crisi è tutt'altro che finita e l'Italia rischia di arrivare esausta al prossimo autunno senza una decisa inversione di rotta. Di fatto, stiamo assistendo passivi ad una falcidie di piccole e medie imprese, con una preoccupante ondata di tagli di posti di lavoro, che la cassa integrazione da sola non basterà a contrastare se, da un lato, si continuerà a sprecare tempo per l'avvio di vere riforme strutturali e, dall'altro, si continueranno a varare misure estemporanee, compreso l'ultimo decreto-legge anticrisi, che presenta solo pannicelli caldi. Nella nostra proposta di risoluzione diciamo con chiarezza, e chiediamo al Governo di avere il coraggio di accettare la sfida, che in fasi di crisi come questa i conti peggiorano comunque e l'unico modo per migliorarli è far ripartire al più presto l'economia, creando quelle situazioni per cui sostegno al reddito e nuove spese per investimenti siano sostenibili, cioè possano durare per il tempo necessario ad uscire dal *tunnel*; il Governo, e con esso il Paese, rischia di doversi trovare fra qualche mese - e mi rivolgo al rappresentante del Governo - a spendere molto di più di quanto previsto perché, per tassi di disoccupazione a due cifre, i fondi per gli ammortizzatori sociali sono del tutto inadeguati, anche mantenendo le regole attuali, e questo significa che dovrà intervenire in corso d'opera o per chiudere il rubinetto delle erogazioni, oppure per ampliare le dotazioni dei vari fondi, rendendo ancora più distorsivi gli effetti della spesa. Il DPEF, signor Presidente, non propone ciò che veramente servirebbe, una seria indicazione di riforma degli ammortizzatori sociali, mentre la disoccupazione è in aumento dovunque e un gran numero di famiglie riducono gli acquisti non più per motivi precauzionali o per paura, ma perché effettivamente i loro redditi, con la perdita del posto di lavoro, stanno raggiungendo livelli di soglia della povertà. Diventano una risposta truccata le misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento degli ammortizzatori sociali previste dall'ultimo decreto-legge n. 78 del 2009 perché, oltre a non rappresentare risorse aggiuntive, in quanto finanziate attraverso la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione del precedente decreto- legge n. 185 del 2008, non risolvono il problema della massa di lavoratori dipendenti o parasubordinati che non hanno diritto ad alcun trattamento in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro: queste misure consistono semplicemente in un intervento di proroga della possibilità concessa ai lavoratori in cassa integrazione. In tempi di grave emergenza è una risposta truccata anche perché tale misura non è di immediata applicazione: sarà infatti necessario attendere l'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, che disciplini le vere modalità attuative della norma. Non si prevede niente per i lavoratori atipici e addirittura nel decreto-legge n. 78 si annullano risorse già destinate all'attuazione di quell'istituto sperimentale di tutela del reddito, quell'*una tantum* nella misura del 20 per cento del reddito percepito l'anno precedente, per i collaboratori a progetto, mentre si sarebbe dovuto procedere in tutt'altra direzione: prevedere una revisione delle condizioni per accedere a tale beneficio, una sua estensione a tutte le forme di lavoro atipico e un incremento del beneficio, perché attualmente questa *una tantum* è semplicemente una miseria. Il DPEF, signor Presidente, pur dedicando un intero capitolo alla tendenza della spesa pensionistica, anche in questo caso non propone alcun indirizzo al riguardo di una riforma complessiva del sistema pensionistico. La nostra spesa sociale nel suo complesso è pari alla media europea, ma il problema è come noi italiani spendiamo quella parte cospicua del PIL. la questione di fondo che tutte le politiche attive a favore delle donne, dei giovani, delle famiglie, della lotta alla povertà e della disabilità sono finanziate con meno della metà di quanto avviene nel resto dell'Europa. Iniziare a spostare quindi le risorse tra le diverse voci di uno Stato sociale è, anche questa, una riforma strutturale più che mai necessaria in un periodo di crisi. Il DPEF, inoltre, amplifica gli interventi varati dal Governo per il sostegno alle imprese, citando la norma prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 sulla detassazione degli utili reinvestiti. Questo è un altro problema che ha delle similitudini con la detassazione degli straordinari, perché con la detassazione degli utili reinvestiti siamo agli antipodi dei più elementari criteri di incentivazione allo sviluppo. Lo sgravio, infatti, non viene concesso all'imprenditore messo in difficoltà dalla crisi o a chi decide di puntare sulle aree depresse, ma viene dato a chi ottiene un risultato degli utili. Si tratta di una detassazione che avvantaggia le grandi industrie penalizzando le imprese piccole e medie che compongono il già fragile tessuto produttivo del nostro Paese e in particolare il Mezzogiorno, le realtà che avrebbero bisogno di maggiori aiuti. proposta di risoluzione vogliamo affermare con chiarezza anche un altro principio: è possibile contrastare la crisi economica anche attraverso il finanziamento di infrastrutture. L'allegato infrastrutture si configura come un elenco della spesa, con un bancomat dei fondi FAS in via di esaurimento, privo di ogni garanzia, sulla certezza delle risorse e dei tempi di avanzamento sia delle grandi che delle piccole opere. L'esperienza insegna che non basta stanziare solo sulla carta risorse finanziarie ma che, per la realizzazione di opere utili in tempi brevi e con costi certi, va riqualificata la spesa statale con una logica di risultato e con una individuazione precisa delle priorità, degli obiettivi dei diversi programmi con un'esatta definizione degli indicatori per misurarli. Abbiamo visto come nella legge di assestamento del bilancio, cosi come nel DPEF, tra le azioni per contrastare la crisi economica sia stata prevista l'accelerazione dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, anche qui con una forte discriminante per gli enti locali. Il problema principale degli enti locali non è tanto la velocità dei pagamenti, ma il limite posto dal patto di stabilità interno che blocca la spesa e impedisce pagamenti e investimenti. Si vuole così, da un lato, sbloccare la capacità di spesa della struttura statale e, dall'altro, verso gli enti locali si conservano norme che irrigidiscono la gestione del bilancio. Anche qui vi è una situazione paradossale, si propone un obiettivo e si opera in direzione contraria. Anche questa è stata un'altra risposta truccata perché nel nuovo decreto anticrisi il problema viene affrontato in modo insufficiente con una piccola deroga per gli enti locali che consente lo sblocco dei pagamenti per una percentuale soltanto del 2,7 per cento dei residui passivi al 2007.

Se a distanza di pochi giorni dalla presentazione di questo importante documento di programmazione, si è costretti a precipitarsi a dire, su tutta la stampa nazionale, che la questione meridionale è al centro dell'agenda del Governo, allora vuol dire che quell'assenza e quel silenzio avevano un significato ben preciso: la strategia politica del non vedo, non sento, non parlo. parlo. Si sa bene che il problema del Mezzogiorno non è né risolto né in via di risoluzione. Si sa bene che i dati diffusi dalla SVIMEZ lo confermano con desolante chiarezza.

ma organizzatore, serio e autorevole, di cui ha bisogno tutto il Paese. Se il Mezzogiorno resta il principale problema nazionale, non è possibile affrontarlo senza un'azione consapevole e di lunga durata della politica nazionale. Il Governo sinora ha dato una risposta semplice: ha finanziato tutte le misure adottate per fronteggiare la crisi togliendo risorse al Sud (18 miliardi di fondi del FAS sono risorse sottratte al Sud), e poi rinvia ai tempi lunghi e incerti di un federalismo, che appare oggi in questa fase più ideologico che non di sostanza. La crisi non peserà sulle tasche degli italiani, ce lo ha ricordato più volte il ministro Tremonti. Ma la verità - anche su queste considerazioni che sono contenute nella nostra proposta di risoluzione - è che molti cittadini hanno già pagato hanno già pagato con meno soldi per la sicurezza, meno per la scuola, meno per l'università, meno per le povertà, meno per gli investimenti dei Comuni, meno per le infrastrutture al Sud, meno per la formazione professionale.

Signor Presidente, la lettura del Documento di programmazione economico-finanziaria per quanto riguarda il sistema della salute del nostro Paese, mancando totalmente di qualsiasi riferimento alla sanità, è l'immagine esemplificativa di come questo Governo non tenga in alcuna considerazione le politiche di tale comparto. Dalla mancata nomina del Ministro competente in poi, le politiche della salute sono state affrontate unicamente come una partita finanziaria diretta dal Ministero dell'economia. Questa scelta politica è ancora più grave nella situazione di crisi economica in cui ci troviamo, che incide negativamente sulle famiglie e le persone creando ulteriori rischi di emarginazione e disuguaglianza. Questa situazione di crisi dovrebbe invece spingere ad un piano di rilancio e di innovazione di tutto il sistema sanitario, un sistema che, non dimentichiamolo, non produce solo spesa ma anche ricerca e innovazione tecnologica, un comparto produttivo importante che produce ricchezza ed occupazione qualificata. Nel Documento di programmazione economica pensavo fosse logico trovare tradotto in politiche di intervento il contenuto del Libro bianco sul *welfare* del ministro Sacconi. Non condivido il contenuto di questo documento e colgo questa occasione per lasciare agli atti tale mio orientamento. In quel documento il tema della sanità è affrontato partendo dalla paventata e, a suo dire, inevitabile esplosione della spesa sanitaria e l'unico rimedio previsto è quello di far pagare i cittadini. Si prevede di realizzare un secondo pilastro di finanziamento di tipo privato, con il ricorso a mutui ed assicurazioni e per realizzare tale intervento si prevede un mutamento del modello di contrattazione, che metterebbe le varie categorie di lavoratori nelle condizioni di contrattare i livelli di tutela dei bisogni a seconda dell'attività svolta e del ruolo sociale; l'esatto contrario del sistema universalistico che la riforma sanitaria del 1978 ha impostato, riforma che, non dimentichiamolo, ci ha consentito di inserire il nostro Paese a pieno titolo nel sistema europeo di *welfare*. In questi giorni il Governo ha lanciato l'allarme rosso sulla spesa sanitaria. Si è utilizzato, ai fini di giustificare un taglio di risorse per la salute sul 2010 alle Regioni, un debito, quello delle Regioni del Sud, che si è accumulato nel tempo senza alcun intervento fino a quando il Governo Prodi ha impostato la manovra di rientro. Ora, la nostra non è una difesa gratuita delle Regioni, ma c'è l'obbligo della chiarezza. Se leggiamo i dati della Corte dei conti ci accorgiamo che la spesa non è affatto fuori controllo. Basta leggere il rendiconto 2008 che riporta i risultati del conto consolidato della sanità per il 2008 e il 2007 e che certifica che il consuntivo è in valore assoluto migliore delle attese.

del luglio 2008. Inoltre, il peso della spesa sanitaria, nonostante ci sia stata la flessione del PIL, si conferma nei livelli previsti, cioè il 6,9 allora che rispetto a queste valutazioni il Governo debba mettere in campo nuovi strumenti. Ad esempio, mi domando come si farà a determinare i costi standard delle prestazioni, di cui il DPEF parla solo nel capitolo parla solo nel capitolo del federalismo fiscale. Questa può essere una grande occasione per mettere a regime un sistema che renda leggibili e confrontabili tra Regione e Regione i dati che attengono all'efficienza, all'efficacia ed all'appropriatezza delle prestazioni. Abbiamo un Paese diviso in due, signor Presidente, anche per quello che riguarda i servizi sanitari. I diritti sono accessibili in forme diverse a seconda di dove si vive; il federalismo fiscale può accentuare queste differenze ma può anche colmarle, dipende dalle politiche del Governo e dalla capacità di mettere in atto un rapporto vero e reale con le Regioni e superare questo contenzioso che le ha costrette ad abbandonare il tavolo del Governo. Come si fa a produrre in questa direzione, se non a partire da una definizione dei LEA, su cui si è aperto da un anno un forte contenzioso? Non si può pensare di far pagare tutto ai cittadini riducendo i servizi, allungando le liste di attesa, aumentando le tasse e i *ticket*. Bisogna impostare una manovra che investa per ridurre e riqualificare gli ospedali, ridurre l'alta ospedalizzazione attraverso una rete di servizi territoriali, riqualificare il ruolo del medico di famiglia, creare la rete per dare la continuità di cura. Di questo non vi è traccia nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come non vi è traccia del piano nazionale per la prevenzione e del piano di contrasto alla cronicità che l'Europa ci chiede e che sarebbe il vero argine all'aumento della spesa dovuta all'invecchiamemto della popolazione. L'Europa considera la salute una ricchezza dal punto di vista economico, sociale e anche una produttrice di coesione sociale. La mancanza di strategie generali per affrontare la crisi e governare il Paese è ancora più grave nel comparto della salute e, per questo, convintamente, voteremo contro questo atto del Governo. Signor Presidente, gentili membri del Governo, onorevoli colleghi, il Documento di programmazione economico-finanziaria prende le mosse dalla crisi economico-finanziaria che, come tutti sappiamo, è partita dagli Stati Uniti nello scorso anno e si è rapidamente diffusa in tutto il resto del mondo, producendo effetti molto importanti anche sull'economia reale. La crisi si è approfondita all'inizio del 2009 in concomitanza con la più forte contrazione del commercio mondiale dal secondo dopoguerra. L'attività produttiva italiana, con la sua forte propensione all'esportazione e il peso rilevante del settore manifatturiero, ha particolarmente risentito del crollo degli scambi internazionali e della forte riduzione degli investimenti. Le previsioni per l'economia italiana, in un contesto internazionale caratterizzato da un sensibile deterioramento del mercato del lavoro, vedono una riduzione del PIL del 5,2 per cento ma già a partire dal 2010 si dovrebbe assistere a una ripresa, con un aumento del PIL dello 0,5 per cento e ulteriori incrementi del 2 per cento il triennio 2011-2013. Nonostante l'elevata incertezza delle prospettive economiche, sia a livello internazionale che nazionale, questo Documento evidenzia alcuni segnali positivi. Il Governo ritiene infatti che la velocità di peggioramento della congiuntura abbia raggiunto un un massimo nel primo trimestre del 2009 e che attualmente gli indicatori di fiducia segnalino un recupero in diversi settori, pur attestandosi a livelli storicamente modesti. Per questo il Governo intende incoraggiare questi segnali di ripresa continuando a garantire condizioni di stabilità per la finanza pubblica, a dare supporto all'economia e ad assicurare la coesione sociale.

si articola in quattro aree programmatiche estremamente importanti che desidero sottoporre alla vostra attenzione: opere avviate, con disponibilità impegnate pari a 31,6 miliardi di euro; 2. opere deliberate, per un valore pari a 116,8 miliardi di euro; 3. opere in corso di istruttoria presso la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture, pari a circa 39 miliardi di euro; 4. opere proposte dalle regioni ed inserite nelle intese generali quadro. Partiamo per esempio dai Corridoi europei di interesse del nostro Paese. Viene sottolineato come l'Unione europea abbia recentemente fornito, con riferimento a tali progetti, una specifica interpretazione della "dichiarazione di interesse comunitario", in base alla quale le opere stradali, ferroviarie, intermodali sono da considerarsi interventi legati allo sviluppo dell'intera Unione, e non dei singoli Paesi. A questo approccio vanno quindi ricondotti anche i flussi di finanziamento derivanti dall'ultimo bilancio comunitario, che per l'Italia prevede l'assegnazione di 25,6 miliardi di euro a valere sui fondi strutturali 2007-2013, e oltre il 16 per cento dei 6,8 miliardi del bilancio complessivo dedicato alle reti TEN. Va poi considerato che il processo di liberalizzazione del sistema ferroviario non si è sviluppato in questi anni secondo criteri omogenei e con tempi contestuali. Alcuni Paesi, fra i quali l'Italia, hanno applicato integralmente i principi contenuti nelle direttive comunitarie, mentre ciò è avvenuto solo parzialmente in altri Stati membri, determinandosi pertanto, nel territorio europeo, una situazione di non piena rispondenza ai predetti principi. Ne derivano conseguenze negative in termini di qualità dei servizi, e, soprattutto, forti squilibri sul piano della competitività e della concorrenza fra le imprese dei vari Paesi. Occorre quindi procedere, in tutti i Paesi dell'Europa comunitaria, alla piena applicazione delle regole della liberalizzazione, anche in considerazione del difficili prospettive del mercato ferroviario: secondo le più recenti previsioni, nei prossimi anni la rete ferroviaria potrebbe assorbire solo il 9 per cento della domanda complessiva di trasporto. Questa tendenza rischia di accentuare lo spostamento già in atto verso il trasporto su strada, con pesanti conseguenze in termini di congestionamento della rete stradale e di impatto ambientale.

sottolineo come questo DPEF intenda rafforzare i sistemi di trasporto pubblico e come, a tale scopo, la delibera del CIPE del 26 giugno scorso assegni 1.424 milioni di euro, che si aggiungono ai 1.440 già assegnati alle Regioni nel corso del 2008 per i contratti di servizio Trenitalia.

successivo che viene sottolineato con forza nel documento è costituito dall'esigenza di procedere ad un'efficace ed efficiente integrazione delle reti di trasporto. L'obiettivo è quello di assicurare, nel nuovo regime liberalizzato dei trasporti, una struttura intermodale che sia efficiente e collegata con il territorio.

onorevoli senatori, signor Vice ministro, senatore relatore, ancora una volta avete scelto di giocare con i numeri e avete confuso i cittadini, che non riescono più a capire come pensate di risolvere i problemi del Paese. Avete realizzato una manovra di politica fiscale espansiva per 18 miliardi di euro, un punto percentuale del PIL, senza comunicarlo al Paese ed al Parlamento. ne è accorto, *in primis*, il servizio del bilancio del Senato, che nel *dossier* n. 16 di questo mese di luglio ha mostrato la realtà. Infatti, nell'assestamento di bilancio approvato in questa Aula la settimana scorsa, alcune variazioni risultano volte a determinare, in concreto, una politica fiscale espansiva. In particolare, signor Presidente, mi riferisco alle integrazioni, alle autorizzazioni di cassa - pari a circa 18 miliardi - finalizzate, in base alla relazione illustrativa, a smaltire buona parte dei crediti nei confronti delle amministrazioni, utilizzando i residui passivi iscritti in bilancio. Questa manovra è risultata funzionalmente connessa con quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. L'aumento delle autorizzazioni di cassa determina, così, un impatto sui saldi tendenziali, in particolare sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, per l'anno in corso, di cui l'assestamento non fornisce evidenza, essendo questo limitato alle variazioni sul bilancio dello Stato. Siete riusciti in questa operazione in questa operazione perché nel DPEF non vi è traccia di questa manovra espansiva, come si può vedere dalla Tavola 1.1 Tavola 1.1 allegata al DPEF stesso. Ogni DPEF contiene una stima del saldo tendenziale (cioè, al netto della manovra di politica economica) e di quello programmatico (comprendente gli effetti della manovra) per l'anno successivo. Lo scostamento dell'indebitamento programmatico rispetto a quello tendenziale misura l'entità della manovra netta messa in atto dal Governo: risanando i conti, signor Vice ministro, lo scostamento è positivo; se si stanno conducendo politiche antirecessive immettendo nuove risorse nell'economia lo scostamento è negativo; se l'intervento di politica economica è neutro, lo scostamento è nullo.

indicando con ciò un non-intervento di politica fiscale per gli anni fino al 2010. Per non parlare poi di quanto previsto per il 2011, dove lo scostamento previsto è dello 0,4 per cento, o per il 2012 e 2013, ove lo scostamento Eppure, signor relatore, non è così: qui è l'inganno! Nel decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, all'articolo 9, in relazione alla «tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni», avete previsto che «i crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato». signor Vice ministro e signor relatore, il Governo è venuto meno all'obbligo di copertura definito dalla Costituzione, sia perché rimanda la copertura dei crediti resi liquidabili alla legge di assestamento, sia perché evita, nel citato decreto-legge n. 78 del 2009 e nell'assestamento, di quantificarne l'onere; il Governo è venuto altresì meno all'obbligo della trasparenza poiché, in presenza di una vera e propria componente di politica discrezionale (18 miliardi di autorizzazioni di cassa finanziati con *deficit*) realizzata con l'assestamento, non ha inserito le previsioni aggiornate di bilancio nel nuovo contesto di programmazione delineato dal DPEF. perché fare una politica fiscale espansiva di questa entità senza renderla pubblica, perché violare le regole di bilancio, perché ingenerare questa confusione degli strumenti, perché aggirare le regole della trasparenza e perché non mettere il Parlamento in grado di conoscere l'operato del Governo. Vi invito a prestare attenzione perché, così facendo, ci mettete davanti ad una deriva autoritaria che si esplica proprio attraverso la politica economica. Nel momento in cui il Governo cela il suo operato al Parlamento, eliminando la possibilità di sedi negoziali e di qualsivoglia controllo, allora agisce al di fuori del quadro democratico in una deriva, che può essere - appunto - di tipo autoritario. Invece di fare la manovra tramite DPEF l'avete fatta tramite assestamento, in totale assenza di trasparenza. Da qui nasce l'impossibilità del Parlamento, cioè della maggioranza e dell'opposizione (e non soltanto dell'opposizione), di intervenire nella formazione della manovra operata del Governo. A questo si aggiunge un'altra questione ancora in ombra: l'aumento della spesa primaria corrente, come accennato dal senatore Morando.

che uno sfondamento di queste dimensioni, così elevato, tanto da essere equivalente ad una manovra di politica economica non sia stato presentato al Parlamento nelle forme dovute.

di fronte alla caduta degli investimenti ed in presenza di una diminuzione del peso degli interessi sul debito pubblico per effetto della caduta dei tassi di interesse internazionali. Il DPEF non riporta informazioni sui livelli e sulla composizione delle entrate e delle spese. L'assenza di queste informazioni rende difficile valutare la politica di bilancio delineata nel DPEF. È questo che vuole il Governo? Agire nella totale mancanza di trasparenza? innanzitutto che il Governo riferisca in Parlamento attraverso il suo Ministro - il più autorevole, senza offesa per gli altri - circa gli effetti finanziari associati all'assestamento, cosa che finora non ha fatto, nemmeno dinanzi alle puntuali sottolineature di questa opposizione, peraltro mai disconosciute dai membri stessi del Governo. Chiediamo che il Governo indichi l'impatto delle misure ivi contenute in termini di fabbisogno e di indebitamento netto e che si assuma pubblicamente la responsabilità politica di aumentare il disavanzo di 18 miliardi di euro. Chiediamo, infine, che dia le motivazioni della scelta allocativa operata, ovvero la scelta di aumentare il *deficit* fiscale di un punto percentuale per pagare i debiti della pubblica amministrazione. La manovra poteva essere fatta anche per altri fini, agevolare le famiglie o i lavoratori, ma il Governo ha scelto di pagare i debiti della pubblica amministrazione. In una democrazia, signor Ministro, il Governo si presenta al Parlamento e motiva le scelte di politica economica. Chiediamo al Governo di ritirare questo DPEF e il disegno di legge di assestamento per ripresentarlo a settembre in un quadro chiaro ed esaustivo dei saldi tendenziali di finanza pubblica. Affinché il Parlamento sia in grado di valutare le stime presentate nel DPEF 2010-2013, è necessario che questi saldi siano stimati al netto degli effetti del disegno di legge di assestamento. L'approccio dell'attuale Governo alla crisi economica, così come rappresentato nel DPEF, signor Ministro, vede consolidata la posizione di un Esecutivo che non vuole prendere alcuna decisione di politica fiscale. È la logica del *wait and see*, senza alcuna strategia organica di rilancio dello sviluppo economico e sociale. In questi mesi difficili i Paesi avanzati hanno affrontato la recessione agendo su quattro versanti: la riattivazione del credito al settore privato; il rafforzamento della rete di protezione sociale; interventi di sostegno della domanda interna (consumi e investimenti); la definizione e l'implementazione di una strategia di prospettiva per rilanciare la crescita economica e sociale. Su tutti questi aspetti la politica economica del Governo italiano è stata debole e attendista, soprattutto in questa drammatica fase di crisi. Con il decreto-legge n. 78 del 2009, così come emerge dai dati del DPEF, si prevede un impiego assolutamente parziale di risorse. Tali risorse si riducono ulteriormente se escludiamo dal calcolo gli interventi destinati ad altri obiettivi (Abruzzo, Alitalia, Fondo per interventi nel settore sanitario, proroga delle missioni di pace, e così via). Al netto di questi obiettivi, signor Presidente, le risorse stanziate in funzione anti-crisi per il 2009 sono 85 milioni di euro. Signor Ministro, nel 2009 avete stanziato 85 milioni di euro, pari allo 0,003 per cento del PIL; nel 2010 volete stanziare lo 0,14 nel 2011 lo 0,15. È inutile che elenchi qui le percentuali di PIL impegnate nei Paesi europei seri ed importanti. Gli effetti di medio-lungo periodo di questo atteggiamento saranno la ridotta capacità competitiva dell'Italia nei confronti del resto del mondo. Mentre gli altri Paesi sono stati in grado di cogliere le opportunità offerte dalla crisi, noi stiamo rimanendo indietro, senza per questo aver migliorato i conti pubblici.

quanto detto dal Governatore della Banca d'Italia in sede di audizione sul DPEF, perché è a tutti noto. Ma, quando arriverà, signor Ministro, il momento nel quale il Governo prenderà la situazione in mano? Saranno ancora gli eventi a determinare gli atti del Governo (come avvenuto tramite l'assestamento) o sarà piuttosto il Paese a governare la crisi al posto vostro? Non è possibile, non è più possibile che, durante la più grave recessione dal dopoguerra, con manovre di politica economica ad impatto zero, non ci sia alcuna riforma strutturale! Un ultimo scandaloso punto, signor Presidente, è rappresentato da quello che Governo e maggioranza stanno facendo per l'Abruzzo: è stato dedicato un capitolo tra quelli principali a questa Regione. La sostanza ve l'ha detta il governatore Draghi: «Per la parte di tali misure espressamente quantificata, l'impatto sull'indebitamento netto

per l'emergenza Abruzzo. Voi scrivete che servono 2.601 milioni di euro per pagare la rete ferroviaria, ma 2.223 non sono disponibili. Dite che 3.605 milioni di euro servono per la rete stradale ma non ne sono disponibili 3.388, e non mi risponda più su cassa e competenza, signor Ministro, perché non è questa la critica che le stiamo muovendo! Come i terremotati aquilani dovranno pagare la loro ricostruzione, così gli italiani dovranno trovare le risorse per uscire dalla crisi. È lei che ha detto, signor Ministro: «La politica sociale è fatta dall'INPS, ma anche dalle famiglie». Ci chiediamo quanto ancora potrete essere governati dagli eventi, piuttosto che governare gli stessi? vivere di non volere», scriveva Thomas Mann; aspettare che torni la ripresa e che tutto si aggiusti da solo è una politica miope che l'Italia non può permettersi, perché nel frattempo, signor Ministro, il sistema produttivo e il sistema Paese nel suo complesso si indeboliranno in modo irreversibile, perdendo competitività con il resto del mondo.

e per chi, come me, ha vissuto, in varie funzioni, i precedenti trenta DPEF non è elemento di eccessivo rammarico e rincrescimento. Abbiamo infatti varato, in quest'Aula del Parlamento, la riforma della legge di contabilità e quindi è sperabile che, dall'anno prossimo, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica coincida, nei tempi e nella coerenza di impostazione della politica economica, con le decisioni concrete che vengono assunte in settembre sulla legge finanziaria. Sta di fatto, però, che in questo Documento di programmazione economico-finanziaria, contrariamente all'opinione espressa da molti senatori dell'opposizione, in realtà c'è un quadro chiarissimo di che cosa è successo negli anni precedenti e di che cosa potrà succedere negli anni a venire.

Troppo spesso questo motto ha due subordinate, entrambe sbagliate: «decidere senza conoscere» e «conoscere senza decidere». Ebbene, signor Presidente, se prendiamo il 2009 come anno spartiacque di quello che è successo negli ultimi anni e di quello che potrà succedere nei prossimi anni,

Il totale della spesa pubblica è passato dal 48,5 al 53 per cento di quest'anno:

Il totale delle entrate pubbliche è passato dal 44,2 al 47,5

lordo. Un piccolo chiarimento rivolto al senatore Legnini: questo è il dato relativo al totale delle entrate e questi sono i dati scritti nel DPEF.

questi dati dimostrano ciò che è successo negli ultimi anni, a partire dal 2006. Il tema che pongo all'attenzione dei colleghi è che, come noto, ogni aumento del peso dello Stato nell'economia, sia sul fronte della spesa che sul fronte delle entrate, quindi anche a parità di *deficit*

circa 1-1,2 punti di crescita potenziale per i prossimi anni, indipendentemente dalla crisi internazionale e dal ciclo economico. Questo è il dato di fatto rispetto al quale è passato il testimone dal Governo di centrosinistra al Governo di centrodestra. Questo è il testimone economico, ma anche politico, che ha avuto in mano questo Governo sin dal suo nascere, ed esso proietta le condizioni e i vincoli per i prossimi anni. Questo è quanto è successo. successo. Sempre assumendo il 2009 come spartiacque, vediamo cosa il DPEF dice che potrà succedere nei prossimi anni.

viene ridotto leggermente, ma rimane attestato attorno al 47 per cento, con una pressione fiscale che resta intorno al 43 di difficoltà dei saldi di finanza pubblica, nonostante si sconti una ripresa dell'economia (che è a «V» negli Stati Uniti e in Cina, ma purtroppo è a «L» in un'Europa che dorme),

Certamente, in un Paese con questo indebitamento, il «rischio tassi» può aggiungere ulteriori elementi questo è quello che il DPEF dice su quanto potrà accadere nei prossimi anni, assumendosi la responsabilità di farlo con grande chiarezza di dati e di numeri e con grande impegno politico. Pongo allora un problema, signor Presidente, signori membri del Governo, onorevoli colleghi. Mi rifaccio a quanto correttamente detto dal relatore di maggioranza, il collega senatore il problema è come rientrare dall'eccesso di spesa e dall'eccesso di pressione fiscale, causato negli anni 2006-2008 dal precedente Governo di centrosinistra, in una situazione economica di gravissima crisi. Questa è la sfida politica che abbiamo tutti di fronte e che ha di fronte il nostro Governo nei prossimi mesi. Si è detto correttamente che occorre ridurre il totale della spesa corrente primaria, si è detto correttamente che occorre ridurre la pressione fiscale, si è detto correttamente che lo strumento strutturale è quello del federalismo fiscale. Ma sappiamo tutti che il federalismo fiscale otterrà questi obiettivi soltanto quando sarà pienamente operativo, cioè tra quattro o cinque anni. E, come giustamente ha sottolineato il collega Garavaglia, c'è il problema di cosa fare, a partire da settembre, per i prossimi due o tre anni, sia in termini di correzione della spesa corrente primaria, sia in termini di riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese.

Mi permetto di ricordare che, quando il collega Morando dice che occorrerà tendere ad una pressione fiscale del 40 dice che occorre tornare alla pressione fiscale che il Governo di centrodestra aveva lasciato nel 2006. Allora, quando il

qualche mese fa, magari tremando, egli ha spinto il pulsante per sostenere i provvedimenti che hanno portato la pressione fiscale dal 40 al 43,5

della mia replica, anche perché non c'è nel merito molto da replicare. Il dibattito non ha infatti risposto a nessuno degli interrogativi, dei rilievi e delle domande che incombono sull'immediato futuro e su quello a medio e lungo termine della nostra economia e dei nostri conti pubblici. Nessuna parola è stata spesa sulle nostre ragionevoli proposte, formalizzate nella proposta di risoluzione che abbiamo presentato. siamo di fronte ad un disastro senza precedenti dei conti pubblici. Non è un giudizio: è un dato di fatto inoppugnabile. Vi sono 10 punti in più di debito pubblico, debito che si attesta intorno al

la spesa corrente primaria fa un balzo del 3 per cento ed è fuori controllo. Eppure siamo di fronte ad un DPEF che omette di indicare una strategia per uscire dal pantano della crisi e dalla voragine che si è determinata nei conti pubblici. Un Governo che dichiara - come ha ricordato ieri il collega Morando che non c'è nulla da fare, aspettiamo che passi, che rinuncia e che non indica una rotta è un Governo che non ha fiducia nelle sue forze e in quelle del Paese. È un Governo che registra e e rinuncia: è questa la vera chiave di lettura della politica economica del Governo di fronte alla più grande recessione dal dopoguerra ad oggi. C'è di più, signor Ministro. Dal luglio 2008 al luglio 2009 abbiamo assistito a un sistematico stravolgimento delle regole che governano la sessione di bilancio, prima della riforma, che pure abbiamo condiviso.

a registrare le scelte fatte in quei nove minuti. Successivamente sono state fatte cinque o sei minifinanziarie *omnibus*. Altro che assalto alla diligenza, abbiamo assistito all'assalto ad un intero convoglio! sottolineato, si utilizza l'assestamento per fare una manovra di sforamento di un punto di PIL, senza trasparenza e in violazione delle leggi di contabilità. Infine, si fa un DPEF, quello di quest'anno, senza indicare gli interventi anticrisi e di correzione dei conti per i prossimi tre anni. Non lo diciamo noi: lo dicono - garbatamente, ma lo dicono

che ci sono state proposte. Insomma, due manovre fuori sessione, fuori sacco, fatte in un Consiglio dei ministri - non è difficile immaginare

il DPEF, alla Camera si fa una manovra fuori sessione di bilancio, collegata anticipatamente al DPEF, il che è una novità, prima che il DPEF stesso venga approvato.

Non solo, ma a fronte dei rilevati - e non solo da noi - errori, ingiustizie, norme incostituzionali (rilievi informalmente sottolineati anche dal Quirinale) contenuti in quel decreto-legge, che cosa si fa? La Costituzione, signor Ministro, signor Presidente, com'è noto, prevede la seconda lettura. La Costituzione non è stata ancora cambiata. Il Governo, pur non avendo fatto la riforma dei servizi pubblici locali, fa tutto *in house*, fa tutto a casa sua, ignorando o tentando di ignorare la volontà del Parlamento. Il Senato ha i tempi per apportare le modifiche e noi siamo disponibili ad assecondare le necessità dei tempi che ci sono dati, ma sentiamo dire e leggiamo sui giornali Dice il Governo: ci pensiamo noi a fare la seconda lettura. Questa è la più grande innovazione costituzionale, signor Presidente, altro che dibattito su bicameralismo e monocameralismo! la norma più odiosa per i terremotati in Abruzzo, ovvero si fanno pagare loro le tasse mentre stanno ancora in tenda, mentre sono senza lavoro e senza aziende. nel quale Camera dei deputati approva questa norma, lei, signor Ministro, e il sottosegretario Bertolaso annunciate: cambieremo, ovvero abrogheremo la legge con un'ordinanza di protezione civile. È incredibile, signor Presidente. Che c'entra il pagamento delle imposte con la Protezione civile? È un mistero: che cosa c'entra? Ce lo dovete dire. Si deve cambiare quella norma. Come si possa cambiare o abrogare una norma di legge con un'ordinanza di Protezione civile credo sarà oggetto di studio

il 2 agosto e non possono rimanere due giorni in più a lavorare, vorrà dire che rimarremo noi qui, per qualche giorno ancora, fino a quando il decreto non sarà modificato. Pensateci fateci sapere. E lei, signor Presidente, si faccia garante del rispetto delle prerogative costituzionali del Senato della Repubblica.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il tema oggetto di questa discussione è il Documento di programmazione economico-finanziaria, l'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria

la legge di stabilità, un testo di grande importanza attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. La ragionevole previsione è che davvero questo sia l'ultimo DPEF. Il Documento di programmazione economico-finanziaria si pone sull'asse del tempo come documento che concentra l'attività del Governo nella sua proiezione futura e che riassume l'attività svolta. L'anno scorso il DPEF era il documento iniziale dell'attività di questo Governo e si sviluppava sull'asse del tempo nella proiezione degli anni della legislatura. Questo in esame interviene dopo un anno e contiene il consuntivo delle cose fatte e la proiezione sugli altri anni della legislatura. L'azione di questo Governo fin dall'inizio è stata determinata in funzione della crisi. Nel vecchio Documento di programmazione economico-finanziaria, quello dell'anno scorso, era scritto: una crisi che arriva e si aggrava. Mi permetto di notare che a quell'altezza di tempo nessuno ancora parlava di crisi. È noto che il nostro programma elettorale conteneva la stessa formula: una crisi che arriva e si aggrava. Naturalmente era difficile prevedere quando si sarebbe manifestata, in che forma, per quale importo. La cifra della crisi era comunque già ben definita definita nella proiezione della nostra azione di governo. Tante cose sono passate da allora. Forse ricordate che la previsione dell'altro DPEF era un'inflazione che scompariva e la speculazione che arrivava.

ridotta e la speculazione si è manifestata ed è ancora uno dei fattori di rischio che insistono sulla ripresa. La nostra azione si è concentrata su tre obiettivi fondamentali: la stabilità dei conti pubblici, la coesione sociale, la tenuta del nostro sistema industriale. conti pubblici, la scelta di anticipare a luglio e di proiettare su tre anni la finanziaria si è rivelata una scelta corretta e correttamente reputata in tutte le sedi internazionali. Non è difficile immaginare cosa sarebbe successo se, nell'autunno della crisi finanziaria più intensa, la Repubblica italiana si fosse trovata coi saldi di finanza pubblica aperti,

L'andamento delle entrate è in linea con le previsioni. E l'andamento delle entrate della Repubblica italiana ha una dinamica meno negativa rispetto a quella che si manifesta in tutti gli altri Paesi. Noi possiamo confermare la previsione di tenuta dei conti pubblici della Repubblica italiana dal lato delle entrate. Certamente, se mancano 5 punti di prodotto interno lordo, mancano corrispondentemente le entrate. Ma - ripeto - la dinamica in Italia è meno negativa di quella che si manifesta in tutti gli altri Paesi europei. Dal lato della spesa trovo davvero curioso e non facile da da comprendere il senso dei rilievi: da una parte ti dicono che devi fare più spesa pubblica, dall'altro lato ti dicono che fai troppa spesa pubblica. Credo che una qualche coerenza di analisi debba essere mantenuta, pur nella dialettica politica. Il profilo della nostra spesa pubblica è anch'esso in linea con le nostre previsioni e con i numeri che abbiamo concordato in sede europea. Vi è una scelta di incremento del profilo di spesa sul 2009, ma questo dipende dalla scelta che abbiamo fatto di ridurre in parte (nella parte possibile) la pregressa situazione debitoria in modo da mettere Confermo le nostre previsioni e la correttezza della legge finanziaria triennale che, con il decreto-legge attualmente in discussione, viene semplicemente aggiornata, aggiornata, includendo un anno in più e modificando alcuni profili che sono naturalmente da correggere. Faccio un esempio per tutti: come abbiamo verificato in sede di G8, la Repubblica italiana non aveva pagato i contributi capitali alla *World Bank*; questa voce, che non era nota come voce di addebito nel 2008, deve essere corretta, ed è corretta nel corso del 2009. concerne la coesione sociale, abbiamo concentrato tute le risorse disponibili sugli ammortizzatori sociali.

luogo, la geografia fa la politica. Questo è un Paese che ha 8.000 Comuni. La capacità di assorbimento della crisi in un Paese che non ha grandi metropoli circondate da anelli di periferia in potenziale rivolta, ma 8.000 Comuni e centinaia di medie città, è un fattore di forza e non di debolezza. Il *welfare* italiano non è fatto solo della macchina pubblica, è fatto anche della famiglia, che è oggetto di concentrazione di molti interventi pubblici. Questo è un altro fattore fondamentale. La tenuta sociale italiana è data dall'INPS, ma anche dalla famiglia e ripeto che questo è punto politico fondamentale. Non possiamo dire che questo è un Paese non pacificato. Questo è un Paese dove il contrasto sociale non si è manifestato finora e noi riteniamo che la scelta di concentrare sugli ammortizzatori sociali e su altri interventi sociali il massimo sforzo possibile sia stata la scelta giusta. Abbiamo stabilizzato i conti pubblici. Abbiamo

A differenza di altri Paesi, questo è un Paese che ha ancora un elevatissimo grado di coesione sociale, e noi intendiamo la coesione sociale come un valore civile fondamentale, ma anche come un valore economico fondamentale, perché la tenuta di un sistema è data anche dalla coesione sociale. la tenuta del sistema industriale, è abbastanza evidente cosa è accaduto. La crisi si è manifestata nell'autunno del 2008 nella forma di una caduta globale della fiducia. L'Italia è stata colpita sul punto in cui era più forte, e non più debole: la manifattura. L'Italia ha la seconda manifattura d'Europa. L'impatto della caduta di fiducia sul commercio mondiale si è manifestato anche sull'economia italiana, su un punto che non era di debolezza, ma di forza: la manifattura, la produzione e l'esportazione. Quello che abbiamo fatto e facciamo è tenere aperti i canali del credito alle imprese. Non abbiamo mai aiutato le banche: abbiamo sempre e solo aiutato le imprese, e la nostra azione di governo è stata ed è nel senso di servire al sistema economico, in modo diretto e indiretto, la maggiore quantità possibile di capitali,

sono i tre obiettivi fondamentali. Ci è stato detto che questo Governo non è caratterizzato da un sufficiente impegno sul quadrante delle riforme. Mi permetto di affermare una tesi contraria.

alla riforma del processo civile, al federalismo fiscale. Credo sia fondamentale una riflessione sul federalismo fiscale come riforma delle riforme, il fatto che essa sia stata approvata con un'ampia maggioranza in Parlamento è indicativo della sua cifra politica. Vedete, questo è un Paese che ha metà della sua attività di Governo fuori dal criterio democratico fondamentale: *no* *taxation* *without* *representation*. Questo è un Paese che ha metà dell'azione di governo, non del Governo centrale ma di tutti gli altri governi, fuori dal vincolo democratico fondamentale. si spende più consenso si prende, senza il vincolo democratico fondamentale che è quello fiscale. Questo non significa che tutto il bilancio del governo locale debba o possa essere finanziato da entrate fiscali: basta una percentuale anche marginale, ma è fondamentale un criterio di responsabilità nell'azione dei governi locali. Si tratta di responsabilità politica e anche di moralità civile. Credo che la possibilità di spendere senza dovere rispondere direttamente ai cittadini sia uno dei fattori di degenerazione della vita civile. Dobbiamo fermare in assoluto un processo che non è solo di crescente irresponsabilità, ma anche di crescente amoralità in troppi settori dell'attività politica. Si dice: non avete posto un limite all'azione dei governi locali, dovete liberalizzare e riformare quel settore. È vero e nel decreto-legge è prevista il punto fondamentale è un altro. Se una Provincia può comprare in Borsa una quota di maggioranza o comunque una quota significativa di un'autostrada senza chiedere ai cittadini se vogliono pagare le tasse per realizzare quell'investimento finanziario, pur non entrando nel merito se sia giusto o ingiusto quell'investimento, vi sembra ragionevole che una Provincia possa comprare un'autostrada senza chiedere ai cittadini se intendono pagare le tasse per tale acquisto? Credo che il discorso sui governi locali debba essere fatto sul presupposto fondamentale e democratico della responsabilità fiscale. *(Applausi dal

Su questo credo sia fondamentale l'azione del Governo e della maggioranza, e anche dell'opposizione. Se volete davvero contrastare l'evasione fiscale, serve anche l'azione dei governi locali, essendo questo uno dei differenziali che ci separano dal resto dell'Europa. La strategia delle nostre riforme prosegue: la riforma della pubblica amministrazione avviata dal ministro Brunetta, la riforma delle università (che è in avanzata fase di discussione) la riforma delle pensioni. Nel decreto-legge è prevista una norma che stabilizza, in ragione della base demografica e delle proiezioni demografiche, il sistema delle pensioni italiano.

preferiamo parlare di interventi e di provvedimenti di medio andare), quella non è una norma particolare, speciale: quella è una norma fondamentale per stabilizzare una voce fondamentale della vita civile del Paese e anche dei bilanci pubblici. Incorporando quella modifica che allinea sul profilo demografico il sistema delle pensioni, avremo un sistema di pensioni tra i più stabili d'Europa. È un punto fondamentale anche in una visione di medio periodo. Per queste ragioni, credo che la politica del Governo fatta nell'anno passato, e sintetizzata e proiettata sul prossimo quadriennio, sia la politica giusta. È stato detto che altri Paesi hanno fatto di più. È assolutamente vero: molti Paesi hanno fatto di più,

negli anni recenti la dinamica del *deficit* e del debito italiano è sotto la media europea. Questi sono i numeri che si acquisiscono in Europa. Credo non sia corretto valutare nelle serie storiche quanto accade in un in un Paese ignorando l'andamento del prodotto interno lordo; credo non sia corretto guardare ad un Paese e non avere un'idea di sistema, una comparazione con quanto avviene in altri Paesi.

la crisi ha evidenziato che quella crescita non era il prodotto sostanziale, strutturale, l'effetto delle riforme; quella crescita era prodotta dalla leva e dalla droga del debito, da plusvalori immobiliari inventati, una cascata di fenomeni che a Ovest e a Est del blocco continentale europeo ha prodotto situazioni di crisi drammaticamente evidenti su tutto lo scacchiere. Da Ovest a Est, da Nord a Sud, quanto resiste il vecchio blocco della manifattura della struttura continentale europea? Dall'Islanda alla Spagna, dal Baltico fino ai Balcani, l'area della crisi si manifesta con intensità superiore a quella che si manifesta in Italia e negli altri Paesi del blocco continentale. Ci possono essere e ci sono dei differenziali; ci sono grandi Paesi che hanno una caduta del prodotto interno lordo maggiore della nostra, altri Paesi che hanno una caduta un po' diversa dalla nostra, ma fondamentalmente la grandezza di riferimento costituita costituita dal blocco continentale europeo indica la tenuta del nostro sistema, e in posizioni che relativamente ad altri Paesi sono migliori e non peggiori. Credo che la scelta prudente e razionale di fiducia fatta da questo Governo sia stata giusta. È la scelta che è stata oggetto del consenso nelle ultime tornate elettorali. la scelta che questo Governo intende continuare a fare.

Ci riferiamo ai problemi del Mezzogiorno che oggi stanno tornando all'attenzione della politica. Non vorremmo che si trattasse ancora una volta della ricerca di equilibri tutti politici nell'animazione di una sorta di pendolo che oscilla continuamente tra omissioni e accentuazioni di interesse, magari per sollecitare interventi straordinari che molto spesso vengono proposti nella logica di affidamento a commissari straordinari, vanificando tutti quegli sforzi tesi a rendere duratura e basilare l'azione diretta a modificare le condizioni strutturali all'interno delle quali il Mezzogiorno opera. Con questo emendamento, che riprende il ragionamento contenuto in un nostra specifica proposta di risoluzione, che è agli atti, noi vogliamo riproporre la questione della visione strategica che è necessario costruire e coltivare per il Mezzogiorno d'Italia, ripresentando non la lettura di una questione particolare, relativa ad una singola e specifica area territoriale, ma ponendo il tema del nostro Paese e della sua funzione nello scenario europeo nello scenario europeo e mediterraneo. La questione, che oggi vede ancora più in ritardo tanta parte del Paese, ha a che fare con la qualità della politica, con il rigore nella selezione dell'allocazione delle risorse pubbliche, con la qualità delle classi dirigenti e con i principi di responsabilità che devono essere praticati. Noi pensiamo che sia indispensabile promuovere un'azione tesa ad ad animare i principi della programmazione, a costruire un percorso in grado di verificare i risultati conseguiti, ad agire perché vengano esaltati i principi di protagonismo e di responsabilità. Se ci fermiamo a riflettere ci rendiamo conto che la questione del Fondo aree sottoutilizzate non si pone soltanto, come tanti colleghi hanno avuto modo di dire del dibattito, in termini di riduzione delle risorse già assegnate e preallocate per interventi nel Mezzogiorno. Il *vulnus* è ancora più profondo perché, di fatto, è stata destrutturata ed impedita un'idea che presiedeva alla nuova fase delle politiche di coesione nel nostro Paese, riferite al ciclo di programmazione 2007-2013. Si era finalmente compreso, in sede nazionale e in sede locale, quanto fosse necessario costruire programmi unitari, di respiro strategico, per superare i ritardi e di come potesse risultare proficuo e importante mettere a disposizione di tali programmi tutte le risorse, quelle di derivazione comunitaria, quelle straordinarie nazionali e quelle ordinarie nella disponibilità di ciascuno degli attori: lo Stato, le amministrazioni centrali, i governi regionali, gli enti locali. Con la legge finanziaria per il 2007 non erano state garantite solo le risorse per il Mezzogiorno e per le aree sottoutilizzate per il ciclo 2007-2013, ma si affermava il principio che rendeva impegnabili, e quindi giuridicamente disponibili, quelle risorse per l'intero ciclo. Ciò al fine di premiare le visioni strategiche e gli investimenti di medio e lungo termine rispetto ad un'azione che oscilla continuamente tra ottusità centralistica e inconcludenza localistica, magari dettata dall'esigenza di non perdere risorse pubbliche assegnate o dalla volontà di fare perché perché comunque fare è meglio che non fare. Con quella impostazione si volevano costruire le condizioni perché il fare rispondesse ad obiettivi condivisi e rilevanti e perché si agisse

situazioni di monopolio o di privativa da parte di taluni soggetti e nelle quali i mercati non esistono anche in ragione della illegalità diffusa e dei poteri criminali stratificati che replicano se stessi. In una situazione di quel genere non servono solo risorse finanziarie aggiuntive ma serve, innanzi tutto, uno sforzo perché lo standard qualitativo nelle attività ordinarie risulti performante, risulti comparabile con gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei servizi, in ossequio ai principi di competitività

serve quanto meno a limitare i danni derivanti da una dissipazione delle risorse e dalla negazione del principio della programmazione per obiettivi,

può essere vinta soltanto se gli investimenti, l'attenzione e la cura del capitale sociale risulteranno in grado di garantire quel recupero di efficienza e di efficacia che le azioni straordinarie eludono, giacché pongono al primo posto il raggiungimento del risultato puntuale piuttosto

La nostra preoccupazione è che la questione meridionale possa in qualche misura risultare assimilata alla condizione di chi vive la malattia come una condizione necessaria, peraltro con la paura di doversene privare. Un Paese moderno deve rinunciare alle azioni estemporanee; deve rinunciare anche al risultato di breve periodo per sostenere quegli investimenti necessari a ridare dignità e protagonismo ai tanti soggetti che, tra mille difficoltà, ogni giorno producono sforzi straordinari per restituire onore, dignità e rispettabilità alle azioni prodotte nel Mezzogiorno. Per tale motivo, presentiamo l'emendamento 4.1, con il quale riproponiamo al centro dell'attenzione l'impegno ad agire affinché la discrezionalità venga limitata, l'impiego di risorse pubbliche possa essere verificato e misurato in relazione all'efficacia e si possa riassumere la priorità delle grandi questioni - la legalità, la lotta alla criminalità e all'emarginazione sociale - ponendo una particolare attenzione, in questo momento di grave crisi economica, al fatto che in modo virulento i fenomeni legati alle estorsioni e all'usura. Noi siamo convinti che tutto ciò si possa fare; siamo convinti che serva al Paese

possa riassumere tale priorità per il bene della collettività nazionale e per garantire un futuro alle nuove generazioni meridionali.

*(Misto-IS)*. Signor Presidente, rispetto a queste tematiche i miei colleghi meridionali partecipano a tanti incontri e a tanti tavoli verdi, assicurando agli agricoltori che interverranno in Parlamento; ma poi in Parlamento, invece, siamo disattenti o votiamo contro il Mezzogiorno d'Italia. È tutto regolare, rientra

di quanto avrebbero dovuto pagare, e ritengo che per un fatto di giustizia ed equità dovrebbero avere il rimborso da parte delle banche delle somme erogate in più. Quanto all'emendamento 4.6, in esso riprendiamo il tema della ristrutturazione

delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei riguardi della previdenza sociale.

Quindi tento di andare avanti, illustrando l'emendamento 4.3, con il quale non si chiede, anche in questo caso, di intervenire con misure assistenziali. Siamo un po' stufi, signor Presidente, di continuare a sentire che, come ricordo perfettamente,

della copertura della cassa integrazione, ma solo ed esclusivamente delle grandi aziende del Nord. L'emendamento 4.3 si rivolge alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno d'Italia, cioè quelle che operano nell'Obiettivo convergenza, che si chiama convergenza perché dovrebbe far convergere i vari fondi per le aree sottosviluppate messi a disposizione dal Governo nazionale, ammesso che lo voglia ancora fare.

di confinanziamento al Mezzogiorno - che consentono di utilizzare i fondi comunitari. Ebbene, per le piccole e medie imprese stiamo semplicemente chiedendo

Se dovessi essere pesante nelle espressioni, direi che nella legge sul federalismo fiscale, la peggiore legge che si potesse realizzare senza aver messo mano al federalismo istituzionale, si afferma che si dovrebbe che si dovrebbe procedere alla perequazione infrastrutturale. Nel frattempo, c'è qualcuno che si è attivato per porre in essere i decreti attuativi sul federalismo fiscale nell'arco complessivo di 24 mesi. Gradirei sapere se delle pari opportunità in Italia dobbiamo continuare a parlare, retoricamente, soltanto per le donne, o se per caso, in tema di un'Italia impostata in maniera corretta sul federalismo, non vogliamo cominciare a parlare delle pari opportunità per i territori: e le pari opportunità per i territori si possono conseguire soltanto se i territori sono messi sulla stessa linea di partenza. Noi meridionali non vogliamo niente di più che assumerci le responsabilità in un'Italia che vogliamo sia realizzata attraverso il federalismo, e quindi la responsabilità delle assunzioni politiche, gestionali e amministrative sui territori, ma non vogliamo essere penalizzati da una sottrazione sistematica di somme che ci competono: non ce le ha regalate nessuno, purtroppo siamo ancora aree in ritardo di sviluppo e quei denari sono stati contrattati con l'Europa. Non li potete togliere al Mezzogiorno d'Italia! *(Applausi dai Gruppi che il presidente Berlusconi troverà 18 miliardi: i 18 miliardi sono quelli che già sono stati sottratti alle aree del Mezzogiorno. Anzi, mentre svolgevamo la campagna elettorale, sui 18 miliardi sottratti ne sono stati sottratti altri 4, e siamo arrivati a quota

prima di mettere mano ai decreti attuativi, per dare vita realmente alla perequazione infrastrutturale. Non mi interessa se viene fatta la Lecce-Maglie o altro: mi interessa l'intero Mezzogiorno che - mi scusino gli amici siciliani - non è fatto soltanto di Sicilia, ma di tante Regioni che si sentono Regioni italiane.

tenendo anche presente che, come tradizione, le risoluzioni di Camera e Senato devono essere, se non proprio identiche, almeno sostanzialmente simili e quindi l'introduzione di ulteriori elementi potrebbe turbare questa sorta di equilibrio.

buona e giusta per riflettere sul *gap* infrastrutturale e per cercare di ovviarlo, con un piano concreto e non con mere rivendicazioni, che senza un concreto allacciamento ad un'indicazione delle infrastrutture potrebbero Tra l'altro faccio presente che l'infrastruttura principale, il Corridoio europeo Berlino-Palermo, è tra le priorità di questo Governo e che il finanziamento delle opere più importanti relative a tale collegamento è stato previsto e verrà

Non vi è dubbio infatti che scendere in particolari così giustamente circoscritti, in un documento che imposta la politica macro e la politica generale del Governo, è un un po' fuori luogo rispetto all'economia dei nostri lavori. Se dovessimo scendere in particolari per tutti gli altri campi, oltre che per quello agricolo, non si avrebbe più un documento di indirizzo sui livelli macro della spesa e delle entrate pubbliche, ma entreremmo nella

Presidente, raccomando all'Aula e ai colleghi della maggioranza l'approvazione dell'emendamento 4.1, che si fonda essenzialmente su una valutazione che non mi pare rispecchiata in alcun modo

Io credo che uno dei temi più significativi dello sviluppo delle politiche di pari opportunità sia esattamente quello di non considerare l'oggetto di tali politiche come un oggetto come un oggetto aggiunto, parziale, marginale, bensì di valutarne l'importanza ai fini complessivi della questione, che in questo caso è quella dello sviluppo dell'Italia, della sua coesione nazionale e della competitività dell'intero sistema Paese.

di capitoli indispensabili per poter attribuire anche al sistema del Mezzogiorno una sua competitività e per consentire ad esso il raggiungimento di quella soglia di cui parlava la senatrice Poli Bortone. Vi è poi la necessità che la cabina di regia coordini e condivida tutte le iniziative di sblocco delle risorse FAS destinate ai piani di sviluppo e di investimento regionali. Ancora, certo, le incentivazioni per le attività produttive localizzate nelle aree svantaggiate e quelle misure di assistenza tecnica, di premialità e di assecondamento, per così dire, per permettere alle amministrazioni pubbliche, non soltanto statali ma anche regionali e locali, impegnate nel Mezzogiorno, impegnate nel Mezzogiorno, di innalzare la qualità dei servizi offerti, di raggiungere quegli obiettivi di servizio nel campo delle funzioni pubbliche essenziali e di rendere più competitive, sotto il profilo dei costi, le prestazioni. Vi è inoltre la necessità di focalizzare interventi e risorse con un'attività di monitoraggio su alcuni obiettivi specifici. Ne abbiamo già parlato - vorrei ricordare solo quest'ultima problematica - quando è stata affrontata in Aula con una mozione del mio Gruppo la questione delle infrastrutture nel Mezzogiorno. Lasciatemelo dire: l'intervento della maggioranza non fu di particolare profondità. Noi torniamo ad evidenziare quelle questioni: corridoio europeo Berlino-Palermo; Alta velocità ferroviaria Napoli-Bari; completamento della della Salerno-Reggio Calabria e ammodernamento degli altri assi, cioè la Statale Jonica e la Carlo Felice; potenziamento del sistema di trasporto locale delle grandi aree urbane meridionali.

fare in modo che i mezzogiorni d'Italia, (per dirla con la senatrice Poli Bortone) siano in grado di rendere più forte e più competitivo il nostro Paese. lo ribadisco, se davvero vogliamo, alla fine della crisi, trovare in piedi l'intero Paese e non assistere ad una desertificazione di metà dell'Italia.

questa mattina in sede di discussione generale. Non vorrei neanche tediare i miei colleghi, anche perché comincio ad essere soddisfatto da grillo parlante, isolato e qualche volta deriso, quantomeno dagli sguardi, in quest'Aula, sollevavo le questioni che riguardavano il Sud, il disimpegno del Governo, nonché la sistematica sottrazione (che oggi il senatore Vegas definisce generoso trasferimento) di risorse dalle aree meridionali verso quelle più ricche del Paese in una fase di grave crisi. Io ho usato termini un po' più brutali ma apprezzo quest'espressione così gentile, purché sia chiaro il senso!

che si abbandonava una scelta fondamentale quale quella del recupero del divario perché ve n'era una più emergente, cioè la salvaguardia del sistema economico-sociale del Paese e della parte

determinazione che un movimento territoriale deve avere rispetto ai temi delle sue comunità, ha sortito un effetto: oggi il tema è all'attenzione del Parlamento ed anche,

che tale percezione si traduca in iniziativa concreta, in scelte precise. E noi alcune scelte precise le abbiamo indicate. Quando cortesemente l'onorevole Vegas ci ha detto che sarebbe stato possibile... *(Il

abbiamo prodotto delle ipotesi concrete, non delle affermazioni assolutamente generiche,

Mezzogiorno desta in me ironia. La frase che essa riporta: «con riferimento al Mezzogiorno, il Governo ha avviato una riforma delle procedure di spesa relative ai fondi destinati alle regioni meridionali, sottoutilizzate), al fine di accelerare la spesa e di assicurare la realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno» è francamente imbarazzante. Il Governo non ha modificato

spostato le risorse dalle aree meridionali più deboli alle aree forti del Paese, in ragione di una strana solidarietà: un Robin Hood alla rovescia. Lo abbiamo sempre detto; oggi ci è stato confermato solennemente in quest'Aula che questa è stata la scelta del Governo, che non possiamo condividere, per cui chiediamo di votare il nostro emendamento 4.8, che contiene misure precise per lo sviluppo del Sud.

perché non abbiamo presentato emendamenti e perché ci sembra un po' surreale questa nicchia di dibattito sull'ultimo DPEF della storia di questa Repubblica.

che il Movimento per le Autonomie voti contro il DPEF. Credo che ciò sia coerente con quanto insieme stiamo dicendo in questo Parlamento.

**Il Senato non approva.**